6 luglio 2011 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze*: «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»

Presidente, colleghi, il provvedimento che oggi richiede l'ennesima fiducia per poter avere una maggioranza che lo approvi è stato presuntuosamente presentato come decreto per lo sviluppo, dunque si attendevano, nell'ambito dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelte coraggiose e innovative. La Germania, infatti, all'inizio della crisi investì 10 miliardi di euro in nuove risorse per università e ricerca, perché riteneva che quella fosse la strada più opportuna per la ripresa economica. Forse, qualche riflessione *a posteriori* dovrebbero farla i nostri Ministri e il Governo. Invece, oggi assistiamo all'ennesimo deludente atto legislativo che, peraltro abbinato all'articolo 19 dell'imminente manovra, concorre a stabilire nuovi tagli, riduzione di personale e servizi. Infatti, riguardo all'articolo 1, relativo al credito d'imposta per la ricerca scientifica, appare assolutamente inadeguata la disposizione relativa al sistema di calcolo solo sulla parte incrementale delle somme destinate alla ricerca, mentre sarebbe stato opportuno, al fine di premiare le imprese che si sono impegnate costantemente nella ricerca, disporre il credito, come aveva previsto il Governo Prodi, su una quota fissa delle risorse investite, indipendentemente dall'ammontare e dall'eventuale incremento. Per consentire poi agli enti di ricerca di poter rispondere alle esigenze di innovazione espresse dall'impresa finanziata, sarebbe necessario rimuovere tutti gli ostacoli alla realizzazione del *turnover* del personale e consentire agli enti medesimi di disporre delle risorse umane necessarie. Tale disponibilità andrebbe garantita anche per le università. Siamo invece all'assurdità di concorsi di assunzione per ricercatori, già banditi da tempo da atenei che rientrano nella soglia del costo del personale del 90 e che non possono più essere effettuati per i tagli successivi a queste risorse. Vorrei solo sottoporre una riflessione: in audizione, martedì scorso, il presidente della CRUI, professor Mancini, ha affermato: «Il contesto finanziario entro cui gli atenei stanno attualmente programmando le assunzioni è obiettivamente assai difficile per il 2011 e addirittura inaccettabile» - sottolineo al Governo: inaccettabile - «per il 2012, con una riduzione del fondo di finanziamento di più del 5 per cento, tale per cui le risorse disponibili allo stato attuale risulterebbero inferiori di gran lunga alle spese fisse sostenute per l'esercizio finanziario di riferimento». Riguardo alla scuola, i commi da 17 a 20 dell'articolo 9 rappresentano nel loro complesso una clamorosa smentita del piano straordinario di assunzione e stabilizzazione del personale precario, insegnanti e ATA, promesso dal Governo prima delle elezioni. L'assenza non solo di tabelle e numeri esatti, ma anche di un impegno chiaro alla copertura di tutti i posti vacanti disponibili, sottolineata da tutte le associazioni professionali e sindacati, è la manifestazione della scarsa capacità della disposizione ad affrontare il problema del precariato. Gli inflessibili richiami alla legge n. 133 del 2008 e al regime autorizzatorio delle nomine fanno peraltro facilmente prevedere la prosecuzione delle assunzioni a contagocce che ha caratterizzato l'ultimo triennio, ben al di sotto della copertura dei posti vacanti e disponibili del *turnover*. La disposizione in questione non può certamente essere motivata come un piano straordinario di assorbimento del precariato ed è totalmente incapace di compensare l'effetto deleterio di quanto previsto dal comma 18 dell'articolo 9, secondo il quale non si applicherebbe alla scuola la norma europea, già recepita nella nostra legislazione, che costringe qualunque azienda, pubblica o privata,

Inoltre, il Governo e il Ministro continuano a mentire quando dichiarano che il piano triennale di tagli di 8,5 miliardi e di 130.000 posti in meno si esaurirà quest'anno, perché andranno a regime nei prossimi tre anni le cosiddette riforme della scuola primaria e superiore, con i relativi tagli di monte ore e relativo personale. Con questa situazione, aggravata dall'articolo 19 della prossima manovra, ci si domanda fino a quando un giovane capace che ambisce a fare il docente dovrà aspettare per entrare in ruolo nella scuola italiana: con il vostro Governo non ne entrerà neppure uno. Altro che politica per i giovani! i giovani! Questo provvedimento reca nel titolo: «Prime disposizioni urgenti per l'economia». Per l'istruzione e l'università di molto urgente c'è da ricostruire la credibilità delle istituzioni, magari con un altro Governo.

oggi la Banca centrale europea - quel mostro giuridico al quale l'Europa ha ceduto una sovranità illimitata, che in democrazia discende dal suffragio universale, e un'ampia autonomia senza chiedere in cambio né regole, né responsabilità, e che tiene sotto scacco la politica e i Governi e si permette, come ha fatto di recente Trichet, di affermare che la Tobin *tax* rappresenterebbe granelli di sabbia all'ingranaggio ben collaudato della speculazione finanziaria, con i derivati e la per alimentare elevati guadagni e *stock option* milionari a misura di banchieri - aumenterà il costo del denaro dello 0,25 per cento, portando il tasso di riferimento all'1,50 rendendo così ancor più complicata la vita di tantissime famiglie indebitate e impoverite anche da tre anni di politica economica di questo Governo. Altro che ministro Tremonti salvatore della Patria! Mentre accade questo, il Governo si accinge a mettere l'ennesima fiducia sul decreto sviluppo, dal titolo ingannevole, forse fraudolento, perché sviluppa solo alcuni interessi, come quello dei banchieri, a danno dei cittadini, delle famiglie, dei contribuenti, soprattutto quelli a reddito fisso, dei pensionati. Questo decreto è indigesto per la maggioranza dei consumatori, ai quali il Governo, specie il ministro Tremonti - che ricorda tanto quel vampiro, quel principe di Valacchia che succhiava il sangue della povera gente - ha ipotecato il futuro, perché, a differenza di quanto aveva affermato in un'audizione alla Commissione finanze del Senato nel novembre del 2008, subito dopo il *crack* della Lehman Brothers, sui banchieri che sbagliano, che dovevano andare in galera oppure essere cacciati, quei banchieri sono tutti a piede libero, eccetto - lo ricordo sempre - il signor Profumo, cacciato dai suoi "compagni di merende" con una liquidazione di 40 milioni di euro. E questi signori banchieri dettano la linea politica a un Governo, il più fedele dei maggiordomi, come è stato dimostrato dal primo atto, quel milleproroghe che ha cancellato consolidate sentenze di Cassazione sull'anatocismo, cancellando i diritti che sono frutto di 20-30 anni di battaglie giudiziarie dei consumatori e della loro associazione. Il secondo atto è rappresentato da questo provvedimento definito come decreto sviluppo appunto perché sviluppa

lo dice l'Italia dei Valori o il senatore Lannutti, cattivo con le banche. Lo dice un giornale, «Il Sole 24 Ore», il giornale della Confindustria,

Il loro potere contrattuale, in un'economia stagnante quale quella italiana, si è talmente rafforzato nei confronti delle istituzioni e della clientela da vederle protagoniste di importanti scelte di politica economica e industriale». ancora Nicola Borzi, un attento giornalista: «le banche italiane alzano il tiro e dettano la revisione delle norme di settore. Il caso più evidente è quello del "decreto sviluppo" che ha rivisto i tassi usurari in senso favorevole agli istituti di credito». A farne le spese - come sempre - è la povera gente: sono gli indebitati, quelli che hanno pagato tassi sui mutui dello 0,50 per cento in più rispetto alla media europea; sono quei cittadini, quegli utenti dei servizi bancari di quel cartello che pagano i costi dei conti correnti (295,66 euro, rispetto ai 114 euro della media europea). E non basta, perché poi il Ministro dell'economia

di reclusione): ebbene, il presidente Vegas, poiché nessuno vuole quelle obbligazioni bancarie, quei 300-400 miliardi di euro di obbligazione, si inventa, come i farmaci da banco, i *bond* da banco, con il bollino blu della massima affidabilità, come quello che le agenzie di *rating* avevano dato a Lehman Brothers, per indurre i vecchi, quelli che si sono sudati il risparmio, a sottoscrivere prodotti bidone. Questo è il secondo atto di questo Governo. Il terzo atto arriverà nella manovra. Lo abbiamo visto con l'inasprimento dei bolli fino al 277 per cento sulla custodia titoli, per penalizzare i piccoli risparmiatori, quelli che si sono sudati 10.000 euro e magari hanno acquistato dei BTP che tengono per cercare, con quelle cedole, di integrare le loro misere pensioni. chi si favorisce? Ve lo siete chiesti? Si favoriscono i conti di deposito, i *family banker* di Mediolanum, i conti di deposito di NG, di Conto Arancio,

che sposta la competenza per le cause di previdenza dai tribunali ai soli capoluoghi di provincia, creando un danno enorme a tutti coloro che devono spostarsi. un bel modo per sviluppare gli interessi delle casse di previdenza, dell'INPS, del presidente Mastrapasqua, che ricopre qualcosa come 54 incarichi: poi si parla della casta della politica, dei costi della politica. Certamente, bisogna ridurre, bisogna dare un esempio. Però, anche un altro senatore ha dimostrato che i costi della politica in Italia non sono molto più elevati rispetto a quelli della media europea. ai metodi vessatori nella riscossione. L'INPS sta inviando, mediante raccomandata con avviso di ritorno, migliaia di ingiunzioni di pagamento, senza peritarsi se tali avvisi siano fondati

«La informiamo che da una verifica dei nostri archivi, risulta che in qualità di rappresentante legale, non ha versato all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti

in caso di mancato versamento, occorre comunicare agli uffici il nome del titolare o del legale rappresentante penalmente responsabile. Ma di cosa parlate! Concludo, signor Presidente, perché

degli italiani, lo si è dimostrato. Continuate a mettere la fiducia, perché i cittadini vi hanno già sfiduciato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, discutiamo l'ennesima fiducia ad un provvedimento del Governo Berlusconi. La fiducia, da ordinaria, è diventata strumento *routine* del percorso legislativo, senza per questo dare vera forza all'attuale Governo, che è ormai ai minimi del consenso nel Paese, e non sarà certo questo decreto che consentirà al centrodestra di risalire la china. Il decreto al nostro esame vorrebbe essere un farmaco d'emergenza per la nostra esangue economia, ma è facile prevedere che non sortirà alcun effetto benefico, soprattutto se associato agli altri micidiali provvedimenti previsti dalla manovra triennale 2012-2014, varata di recente dal ministro Tremonti. Analisti, sindacati, imprenditori hanno chiesto in questi mesi a gran voce misure per la crescita, nella convinzione che anche la meritoria opera di riduzione del debito, come ci chiede l'Europa con il Patto euro euro plus, può avere successo solo con la ripresa forte della nostra economia. La presidente di Confindustria Marcegaglia ha giustamente detto, pochi giorni fa, che crescere dell'l per cento non basta; per creare occupazione occorrono anche gli investimenti, soprattutto in settori come l'edilizia e le infrastrutture, in grado di fare da volano per tutta l'economia. Del resto, Mario Draghi, nella sua ultima relazione come governatore della Banca d'Italia, ha ribadito il medesimo concetto: l'Italia è indietro nella dotazione di infrastrutture rispetto agli altri principali Paesi europei. Non vi sono solo meno investimenti, ma anche - dice Draghi - «incertezza nei programmi, carenza nella valutazione dei progetti e nella selezione delle opere, frammentazione, sovrapposizione di competenze, inadeguatezza delle norme sull'affidamento dei lavori e sulle verifiche degli avanzamenti». Tutto ciò ha come risultato opere meno utili e più costose che altrove. Con il combinato disposto di questo decreto e del prossimo, la situazione sicuramente è destinata a peggiorare, come dirò tra breve. il settore delle costruzioni ha pagato un prezzo pesantissimo alla crisi (oltre 230.000 posti di lavoro in meno, senza contare quelli dell'indotto), mentre non si vede ancora il sereno sul prossimo futuro, se è vero che gli investimenti continuano a calare (meno 6,4 per cento nel 2010, almeno un ulteriore meno 4 per cento è previsto per il corrente anno 2011). Stime e dati dell'ANCE, l'associazione dei costruttori, ci dicono che dal 2008 al 2012 il settore avrà perso in termini reali per cento, tornando così ai livelli del 1994; ripeto, ai livelli del 1994, non del 2004, cioè quasi vent'anni fa: in questo settore stiamo perdendo vent'anni di Di fronte ad un quadro così drammatico, la risposta del Governo è incerta, contraddittoria, incapace di mettere in campo vere misure per il rilancio delle opere pubbliche, piccole e grandi. Ricordo che non solo le grandi opere, ma soprattutto quelle piccole dei tanti Comuni e enti locali sono in grado di dare un ristoro e un impulso vero al rilancio della nostra economia: della nostra economia: oltre il 60 per cento delle opere sono piccole opere, ma mettono in campo tantissime migliaia di imprese. Se da un lato - e questo è un elemento di grande contraddittorietà dei provvedimenti del Governo - nell'articolo 4 del cosiddetto decreto sviluppo si prevede l'estensione del campo di applicazione dell'istituto della finanza di progetto, nella manovra triennale vi sono provvedimenti che certo non incentivano i capitali privati, di cui, lo ricordo, abbiamo un gran bisogno, considerata la scarsità di risorse pubbliche. Vengono cioè penalizzati fiscalmente gli impieghi dei capitali privati nelle opere invece, nel decreto sviluppo si vorrebbero avere più investimenti, essere più attrattivi per i capitali privati. Analogamente, non ci convince la riforma dell'ANAS, che discuteremo nei prossimi giorni. Se qualcuno nel Governo pensa di risolvere il conflitto di interesse dell'ANAS, oggi arbitro e giocatore della partita autostradale, con la ministerializzazione delle funzioni di vigilanza, controllo e programmazione, ebbene costui è fuori strada. Più che a Colbert, Tremonti con questo provvedimento sembra vicino a Breznev e alla Russia sovietica. Al contrario, non serve un provvedimento per trasformare *in house* il lavoro di ANAS: serve un'autorità di regolazione terza, indipendente e forte, non il Ministero. È così facile prevedere che renderete ancora più difficile qualsivoglia politica delle infrastrutture. Se l'Italia si è trasformata nel Paese del non fare, i responsabili siete voi; responsabile è l'assenza della politica del Governo, non i No Tav che bloccano la Val di Susa. Siete voi che avete bloccato tantissimi interventi, perché un conto sono le *performance* del presidente Berlusconi a «Porta a Porta» (vi ricordate quante belle infrastrutture disegnate su quella lavagna!), buone per la campagna elettorale; altra cosa è impegnarsi a far marciare i cantieri. Anche in questo campo avete fallito. Per queste ragioni vi negano la fiducia gli italiani, *in primis* gli imprenditori; per queste ragioni ve la neghiamo noi del Partito Democratico. Grazie colleghi senatori, rappresentanti del Governo, riflettendo sui contenuti del decreto-legge sviluppo e sul mio intervento, ho avuto la certezza sta ripetendo costantemente uno stesso evento e uno stesso percorso; ho avuto il senso dell'assoluta immobilità dell'azione del Governo. A partire dalla cosiddetta finanziaria estiva del 2008, quando il ministro Tremonti, con un colpo a sorpresa, ha innovato tutte le procedure della finanziaria e ha intrapreso la via pesantissima dei tagli agli enti locali (8 miliardi di euro), alla scuola (8 miliardi di euro), all'università (svariati miliardi di euro), alle Regioni, attraverso il taglio alla sanità, ebbene da allora non abbiamo fatto altro che vedere il ripetersi di situazioni sempre uguali a se stesse. I decreti molto spesso prendono dei nomi positivi. È abile il Governo a dare dei nomi positivi, ad esempio questo è il decreto sviluppo, che non rilancia niente affatto l'economia, l'occupazione, appunto lo sviluppo necessario del nostro Paese; nomi che non corrispondono assolutamente ai contenuti di queste norme. Si susseguono poi, con una costanza assoluta, i voti di fiducia, per cui i testi proposti dal Governo sono del tutto blindati, non cambiano per nulla dall'inizio Le manovre finanziarie si alternano poi alle cosiddette leggi *ad personam* e questi sono gli unici atti di cui il Senato discute, anche se non può cambiare nulla. Da ultimo, abbiamo visto il tentativo, peraltro fallito, di inserire una norma *ad aziendam*, cioè *ad personam*, in una manovra finanziaria. L'alternanza tra manovre finanziarie, di cui non condividiamo i contenuti, e leggi *ad personam* è la caratteristica di questa legislatura. Tutti i decreti - anche questa è una costante - sono pieni di norme totalmente diverse le une dalle altre, decreti *omnibus*, ma in tutti c'è una costante: un insieme di norme che tagliano nei settori della scuola, dell'università e della ricerca.

Ne cito alcune. Potrebbe essere positivo aver introdotto il credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca. Lo è sicuramente. A mio avviso, era stato uno degli interventi molto importanti attivati dal Governo Prodi. Ma non è positivo il fatto che il credito d'imposta sia riconosciuto solo per l'incremento delle risorse investite in ricerca, cosicché quelle imprese che hanno investito con continuità, anche negli anni più duri e più difficili, quelle imprese che sanno che la ricerca non è un *spot* ma un'azione di lunga lena, ebbene queste sono totalmente penalizzate mentre le altre, quelle che cominciano adesso proprio in nome di contributi e di incentivi, possono avere forti opportunità. Così non va, perché ancora una volta coloro che sono più seri vengono penalizzati.

che sospende per la scuola la norma europea sulle assunzioni dei precari, quella che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere i precari se questi hanno lavorato per tre anni consecutivi nello stesso posto di lavoro. Dice la norma: ma la scuola ha la specificità dei supplenti. È vero, ma

introdurre, anche nelle norme sulla scuola pubblica, una sostanziale privatizzazione. C'è un disegno evidente di demolizione della scuola pubblica in quanto grande istituzione nazionale che garantisce a tutti i cittadini pari opportunità e pari diritti e che costituisce una leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale

Ministeri, ruoli d'indirizzo e di programmazione propri del MIUR, oltre che di gestione di temi importantissimi per il futuro dei giovani che sono il diritto allo studio e la premialità

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ha davvero un che di paradossale il rito di questa discussione che si ripete e che l'Aula del Senato sta ospitando tra ieri e oggi per la definitiva conversione in legge del cosiddetto decreto sviluppo. Appare lontano il Paese reale, quello delle famiglie che vedono ridursi progressivamente la capacità di spesa; delle imprese i cui livelli di produttività sono ancora molto al di sotto dei livelli pre-crisi; dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e dei giovani che non riescono a trovarlo, come ricordato ancora qualche giorno fa dall'ISTAT. È un Paese che negli ultimi tre anni ha visto drammaticamente aggravarsi il proprio dualismo territoriale tra Nord e Mezzogiorno. Appare anacronistico questo provvedimento salutato due mesi fa come la "scossa" all'economia e rivelatosi del tutto inadeguato e, peraltro, ormai superato da un altro provvedimento d'urgenza, l'ennesimo decreto-legge con cui il Governo ha licenziato nei giorni scorsi la cosiddetta manovra da qui al 2014. Quest'ultima agisce come una mannaia sugli enti locali, sulla sanità, sul *welfare*, che avrà magari la possibilità - ce lo auguriamo - di raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio, come concordato con l'Unione europea, ma che - ne siamo certi senza alcun dubbio avrà da subito un ulteriore pesante effetto depressivo sull'economia reale, spingendo il Paese lungo il crinale della recessione. Proprio per queste ragioni il Paese ha davvero e con urgenza bisogno di interventi capaci di produrre crescita e sviluppo, che siano in grado di rinvigorire e innovare il sistema produttivo e industriale del Paese e rilanciarne i consumi. Di tutto ciò, però, non vi è traccia nel provvedimento che stiamo discutendo. Molti colleghi del mio Gruppo si sono soffermati sulle criticità, le contraddizioni e le scelte errate presenti in questo decreto: vorrei dedicare questi pochi minuti ai contenuti che vi avremmo inserito noi, se Governo e maggioranza, e maggioranza, con maggiore lungimiranza, avessero accolto il nostro invito al confronto di merito e non avessero, ancora una volta, fatto ricorso al perverso binomio che caratterizza il vostro modo di governare e la vostra quotidiana ostilità verso il Parlamento ancora una volta alle prese con un decreto-legge con annesso voto di fiducia, il Abbiamo proposto significative correzioni ai tre articoli relativi al credito d'imposta, al fine di rendere la misura realmente efficace ed esigibile per le imprese: gli investimenti nel Mezzogiorno, prevedendo una copertura finanziaria adeguata per rendere tali disposizioni immediatamente attivabili e non soltanto a seguito dell'autorizzazione in sede comunitaria. In relazione ai vincoli del Patto di stabilità, le nostre proposte intendevano consentire almeno ai Comuni virtuosi di poter liberare dai 2 ai 4 miliardi di euro per opere pubbliche urgenti, quali la messa in sicurezza delle scuole, del territorio o investimenti in ambiente e mobilità sostenibile.

Così come in tema di ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, abbiamo indicato uno strumento concreto per alleggerire il peso che il fenomeno ormai ha assunto ai danni soprattutto delle piccole e medie imprese. Si tratta della istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un fondo finalizzato ad anticipare alle aziende private i crediti da esse vantate nei confronti delle pubbliche amministrazioni; In materia di semplificazione, abbiamo proposto che a cittadini e imprese sia riconosciuto un credito d'imposta sulle spese sostenute per l'adeguamento a eventuali nuovi adempimenti così Non comprendiamo il motivo per cui, mentre la maggioranza saluta alcuni timidi e inefficaci interventi previsti in questo decreto-legge come la rivoluzione del rapporto tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione, nel contempo il Governo, alla chetichella, nel corso dell'esame del disegno di legge sullo statuto delle imprese imprese nella 10a Commissione permanente, presenti emendamenti volti a sopprimere due interi articoli del testo approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, riguardanti la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Abbiamo ancora avanzato proposte precise in materia di efficienza energetica, proponendo la stabilizzazione a regime della misura di incentivazione degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici, ora prorogati al 31 dicembre 2011. Una misura che in soli tre anni ha prodotto 400.000 nuovi interventi e che ha rilanciato il settore dell'edilizia e della piccola e media imprenditoria. Tema di grande attualità e decisivo, quello dell'efficienza energetica, per una moderna e duratura strategia energetica nazionale, come proprio ieri ha autorevolmente richiamato nella sua relazione annuale la stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nel campo delle infrastrutture, nonostante la timida propaganda che vi contraddistingue, la realtà è quella di una spesa pubblica in conto capitale che ha subito nel corso degli ultimi anni tagli consistenti e feroci, che hanno sostanzialmente bloccato la realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche e che stanno restringendo i servizi universali come il trasporto pubblico. Con la fiducia ci impedite di limitare la portata di tali tagli, potendo invece accogliere i nostri emendamenti volti a rifinanziare (e abbiamo trovato le risorse per poterlo fare) gli interventi infrastrutturali nei grandi corridoi ferroviari, nei porti e negli aeroporti, gli interventi per il trasporto pubblico locale e per la manutenzione straordinaria delle strade, la banda larga. Vi è, infine, l'immenso campo delle liberalizzazioni, su cui avete in questi anni tradito non solo le vostre promesse elettorali, ma persino i principi liberali a cui spesso, con scarsa coerenza, vi richiamate. In realtà, ogni iniziativa volta a spostare risorse dalla rendita e dalle posizioni dominanti verso il lavoro e a favorire l'apertura e la trasparenza dei mercati è di per sé una norma capace di produrre ricchezza in questo nostro Paese. Anche questo provvedimento è un'occasione persa. Le nostre proposte, qualora approvate, oltre a non avere oneri a carico del bilancio dello Stato, nel campo delle liberalizzazioni, avrebbero qualificato il provvedimento, con l'effetto immediato di favorire la crescita e di accrescere la concorrenza nell'ambito del settore dei servizi, intaccando i settori tutelati, i privilegi, gli sprechi, con l'obiettivo di produrre effettivi risparmi per imprese e famiglie. Penso al settore dei carburanti, alla separazione proprietaria della rete di trasporto del gas, alla trasparenza dei costi dei servizi bancari, al funzionamento del mercato assicurativo. del mercato assicurativo. Queste sono alcune delle scelte che noi avremmo fatto perché davvero questo decreto meritasse di essere definito sviluppo, perché davvero potesse esserci una "scossa" per l'economia, che avete annunciato ma che è lungi dall'essere intravista dal Paese, e il sistema produttivo ne avrebbe guadagnato. Avete ancora una volta scelto la scorciatoia degli annunci roboanti privi di alcun effetto concreto sulla vita quotidiana di cittadini, famiglie e imprese, mentre il Paese si avvita su se stesso in una continua depressione di cui non si intravede la fine.

provo sempre disagio quando non ritrovo coerenza tra forma e contenuto di un oggetto, quando denominazione e sostanza non coincidono. Fatico ad utilizzare le categorie del giudizio in modo piano, perché ho l'impressione di legittimare una finzione. Questa è la condizione nella quale ci siamo trovati con assoluta costanza dall'inizio della legislatura di fronte alla maggior parte dei provvedimenti economici; questa è la condizione in cui ci troviamo anche oggi, messi ancora una volta - in questo, con assoluta coerenza - di fronte ad una richiesta di fiducia. La gravità della situazione economica e sociale in cui si trova il Paese impone verità, e non si può dichiarare fiducia negli esiti di un provvedimento che prescinda da una valutazione veritiera dei suoi presupposti e della sua fattibilità. L'enormità della sproporzione tra la valutazione della situazione dell'Italia descritta per tre anni e la consistenza delle azioni poste in campo per correggerla è resa autoevidente dai numeri, che svelano la bugia della crisi prima negata, poi assunta a giustificazione di ogni contraddizione ed inerzia. Milioni di disoccupati ed inoccupati, centinaia di migliaia di posti di lavoro persi, migliaia di imprese in *default* o in stallo, senza una prospettiva di ripresa, da un lato; dall'altro, tagli alla spesa indiscriminati e depressivi, riforme economiche sempre rinviate, riforme sociali condotte all'insegna dell'iniquità, con detrimento dei soggetti che da sempre pagano i prezzi più alti: le donne, che non lavorando, lavorano il doppio; i giovani, intrappolati tra disoccupazione e precarietà, le famiglie a basso e medio reddito, sempre più esposte all'isolamento ed alla povertà. È stato detto in quest'Aula: «la nostra lettura della condizione di difficoltà in cui versa il Paese è la stessa; diverse sono le soluzioni proposte». Sbagliata la prima, vera la seconda. Voi leggete un Paese attraverso la condizione di alcuni, ceti o territori che siano, e, a partire da essa, determinate le politiche per molti. Noi cerchiamo di usare, all'opposto, la lente dell'interesse generale e della coesione sociale. Voi definite «moderna e postideologica» ogni scelta che confermi e approfondisca lo squilibrio sociale e la segmentazione degli interessi. In questo senz'altro siamo diversi, perché le nostre proposte vanno in direzione opposta. Questo decreto tradisce se stesso già dal nome. Promette sviluppo e ne segnala, finalmente, l'urgenza, ma propone pochi interventi, di assai dubbia sostenibilità ed efficacia e, per la quasi totalità, ne rinvia l'attuazione a provvedimenti successivi. Allora, delle due l'una: se l'urgenza sussiste, le misure devono essere immediate (e sappiamo quanto siano tardive); se l'urgenza, al contrario, non sussiste, perché un decreto e perché la fiducia? Non lo aiuta, poi, la sua collocazione temporale, che lo vede schiacciato nel dibattito e nei contenuti concreti dall'incombere della manovra di correzione dei conti che, per entità e contenuti, rende assolutamente estemporanea la funzione di questo decreto. Segnalo, a margine, a proposito di coerenza tra forma e sostanza, che il Parlamento discuterà la manovra economica più pesante degli ultimi 20 anni in un tempo all'incirca dimezzato rispetto a quello di discussione di un decreto sostanzialmente inutile. Incoerenza e inefficacia riguardano, purtroppo, anche le misure, pur minimali, che attengono il sostegno all'occupazione. Con il credito d'imposta per le assunzioni al Sud, il Governo riprende, tardivamente, una indicazione delle opposizioni, recuperando provvedimenti già avviati dal precedente Esecutivo. Lo fa, però, in una proporzione non valutabile, non chiarendo effettivamente l'entità delle risorse destinate allo scopo. La consistenza reale di questo intervento è nella sostanza rinviata alla negoziazione in sede europea e ad una decretazione successiva. Ne consegue che si approva una misura di stimolo all'occupazione senza esattamente esattamente conoscerne la concreta e reale portata. Prova ne sia il fatto che, dopo aver insistentemente affermato, nella Commissione di merito, che l'obiezione da noi proposta era priva di consistenza, il Governo ha accolto in Commissione bilancio un ordine del giorno dell'opposizione che lo impegna a rendere certe ed immediatamente attivabili le risorse destinate a finanziare questa misura. I soldi non sono materia virtuale: o ci sono o non ci sono. Decidetevi! Inoltre, l'attuale situazione del mercato del lavoro è caratterizzata da uno stato di segmentazione del tutto particolare, che vede sottorappresentati in via assolutamente prevalente i giovani e delle donne. L'utilizzo di uno strumento di stimolo all'occupazione di tipo tradizionale, che misura lo svantaggio occupazionale con il metro classico della lunga durata dell'assenza dal lavoro, non tiene conto né degli effetti indotti dalla crisi e dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali né, appunto, della segmentazione del mercato del lavoro, che vede soprattutto i giovani presenti con la discontinuità tipica della precarietà oppure non li vede affatto, perché del tutto alieni, per scoraggiamento, dispersione o intrappolamento nel lavoro irregolare, dai meccanismi di rilevazione della disoccupazione. Il provvedimento rischia di non produrre - sempre che venga finanziato - alcun effetto concreto. Non so poi ascrivere ad altro che non sia la pervicace affermazione di una primazia formale - in assenza di un primato sostanziale - da parte della maggioranza di governo, il rifiuto di accogliere la nostra proposta sul credito d'imposta per per le imprese e il lavoro autonomo dei giovani, per poi inserire una misura assolutamente analoga nella manovra di cui discuteremo nei prossimi giorni. Auspico che almeno in quella sede ci si preoccupi di finanziarla adeguatamente. Ma di Ma di promesse negate questo provvedimento è una vera festa. Era stato promesso che il primo provvedimento economico utile sarebbe stato il veicolo per mettere mano a problematiche gravissime, derivanti da precedenti provvedimenti economici del Governo. Ricordo solo il blocco delle Ricordo solo il blocco delle assunzioni, che ha penalizzato 1.800 lavoratori somministratati dell'INPS, che ancora attendono che si attui il dispositivo di una risoluzione approvata a marzo alla Camera, e la

Ma, come d'uso, la beffa peggiore riguarda le donne. Qui, davvero, lettura dei problemi e soluzioni proposte non potrebbero essere più diverse tra maggioranza e opposizione. Nonostante in tutte le sedi politiche ed economiche più autorevoli, dalla Commissione europea a Bankitalia, si affermi che le azioni in favore dell'occupazione delle donne e le politiche per lo sviluppo sono intimamente correlate, essendo le prime di stimolo e di traino per il secondo, il decreto sviluppo ignora completamente le donne. Di più, diventa estemporaneamente il tramite del loro scherno, allorquando qualche giorno fa il ministro Sacconi, messo alle strette in quest'Aula, durante il *question time*, sullo scippo delle risorse derivanti dall'aumento dell'età pensionabile delle donne del pubblico impiego, millantava un fantomatico emendamento al decreto sviluppo che avrebbe restituito le risorse sottratte al fondo per la conciliazione e alle politiche per la famiglia. Una clamorosa bugia! Non solo non c'è, né c'è mai stato, nessun emendamento della maggioranza o del Governo al decreto, ma lo scippo è confermato all'articolo 13 della manovra, e lo sarà per i prossimi 10 anni. Migliaia di donne lo stanno denunciando, le stesse che hanno denunciato il 13 febbraio scorso l'insostenibilità di una cultura e di una politica di governo ipocrita, paternalista ed autoritaria, che negando la soggettività delle donne nega all'Italia la civiltà e il futuro. Lo stanno denunciando le stesse donne donne che vi hanno bocciato nelle ultime urne e che vi manderanno a casa, se solo riusciremo ad andare a votare. è da tempo ormai che dentro e fuori quest'Aula è maturata una profonda convinzione: questo Paese ha bisogno di sviluppo; è necessario, direi indispensabile, investire sullo sviluppo.

L'ISTAT ci fotografa un Paese che continua a non crescere, mentre altri Paesi europei hanno agganciato la ripresa, come dati ormai noti ci dicono. L'Italia purtroppo presenta tre primati negativi: non cresce, non aumenta l'occupazione, non si sviluppa. È ferma. Le statistiche ci presentano condizioni di vita diffuse per gran parte delle famiglie italiane che non migliorano, anzi, per alcune fasce di popolazione si aggravano e per alcune aree territoriali sono divenute insostenibili. Penso a gran parte del Sud del Paese, dove i tassi di inattività e le cifre della disoccupazione sono in generale preoccupanti e quelli della disoccupazione giovanile allarmanti al limite delle speranze di prospettiva per un Paese sviluppato di questa parte del mondo. Cifre da collasso che sfiorano il 40 per cento della disoccupazione giovanile e femminile. Di questo, forse, si doveva occupare, almeno in parte, un decreto sullo sviluppo? I disoccupati sono appunto giovani, donne, in particolare del Mezzogiorno. Il lavoro non dovrebbe essere la principale assillante preoccupazione di questo Governo, visto che esso è la principale assillante preoccupazione del popolo italiano? È forse pensando di rispondere in parte a questi quesiti - ma non ci siete riusciti - che avete annunciato con grande enfasi alcune misure: il credito d'imposta sulla ricerca, il credito d'imposta per le aree meridionali per favorire occupazione e investimenti, che si svelano però nella loro vera funzione di *spot* pubblicitari. Vediamo il perché. Il credito d'imposta sulla ricerca, pari al 90 per cento, sembra davvero una misura opportuna, ma - e qui si scopre la finzione - esso è da calcolare sulla spesa incrementale, cioè sulla differenza di spesa tra questo anno e gli anni precedenti. In sostanza, bene che vada, esso si riduce in realtà al 10-12 per cento, anche perché come è ben noto, è proprio in questi ultimi anni che la spesa sulla ricerca è stata drasticamente tagliata da questo Governo con la nostra più ferma opposizione, confortata anche dalle esperienze di altri Paesi europei che, nonostante la crisi e la durezza delle manovre, hanno scelto di investire sulla ricerca. Inoltre, questa misura appare, oltre che modestissima, assolutamente non attuale, perché subordinata - come già evidenziato rispetto al credito d'imposta dalla senatrice Ghedini - all'approvazione da parte della Commissione europea, spendibile prevedibilmente tra 18 mesi. Altro che scossa all'economia! Questa maggioranza, sfuggendo ad un vero confronto nell'interesse del Paese, e non da ora, ma da sempre, forte del principio dei suoi numeri, ma non delle sue idee, ha proposto solo tagli lineari indifferenziati in tutti i campi, senza aggredire il nodo delle riforme. I tagli lineari e ragionieristici si sono dimostrati prevalentemente iniqui, improduttivi e incapaci di ridurre le cause strutturali dell'aumento della spesa pubblica. Veniamo ancora ad un altro esempio delle misure contenute nel provvedimento: il credito di imposta per l'occupazione e il credito di imposta per gli investimenti nel Sud. Sud. Naturalmente sono misure da noi condivise e non potremmo che essere d'accordo; si tratta di misure utilizzate da tempo - ripeto: da tempo - dai Governi di centrosinistra, che hanno fatto di più, utilizzando anche il credito d'imposta differenziato per favorire l'occupazione femminile nel Mezzogiorno. Eppure, quando nei mesi scorsi abbiamo avanzato queste proposte, esse sono state respinte; oggi vengono sbandierate, ricorrendo alla metafora della sferzata, mentre non contengono alcuna operatività, ancora fumo. Se ci aveste ascoltato, oggi sarebbero già operative. Ora invece non lo sono; anch'esse sono infatti soggette alla negoziazione della Commissione europea. Grazie ai nostri emendamenti una di queste misure, in attesa dell'autorizzazione, potrà forse diventare operativa attraverso l'uso dei fondi FAS. Ma c'è da chiedersi, ancora e inoltre: dove sono le opere pubbliche disponibili che il CIPE ha bloccato? Dove avete esercitato quella capacità di governo e di *governance* che sarebbe stata necessaria per ristrutturare in parte l'utilizzo dei fondi europei nel Mezzogiorno, sia per quanto riguarda i PON, sia, attraverso una giusta concertazione, per quanto attiene ai POR? Dov'è il fantomatico piano per il Sud? Certo, ciò richiedeva concertazione, fatica, vincere resistenze ministeriali e regionali, ma era sicuramente una strada da perseguire in modo autorevole, per utilizzare risorse in modo più efficace, sinergico, indispensabile per superare i *gap* strutturali nel Mezzogiorno del Paese. Ma l'arte del governo è cosa complessa e non coincide, se non in piccola parte, anzi talvolta perfino contrasta, con l'arte del comando, che fino a che avete potuto è stata la sola capacità e abilità che avete dimostrato. È difficile seguire il dibattito di questa maggioranza, sia in questo decreto, sia in generale sulle proposte per lo sviluppo economico del Paese; è un susseguirsi di proclami, dichiarazioni, promesse, non scelte, senza un'analisi realistica che vada nel profondo, che richieda esercizio del governo*,* coraggio di scegliere e di selezionare investimenti e priorità, tagli e risorse. Siamo invece di fronte all'ennesimo provvedimento di tipo elettorale, varato nel pieno della campagna per le amministrative, che non è servito a nulla, visti i risultati; un decreto fatto in fretta, senza risorse aggiuntive e senza una strategia per la ripresa e per l'occupazione. Su questo provvedimento si profilano già le ombre di una manovra di correzione dei conti pubblici che appare insostenibile: manovra doverosa e necessaria per gli impegni europei, ma - ripeto - insostenibile per il suo contenuto. Volete continuare ancora con i tagli lineari, nonostante lo stesso governatore Draghi abbia detto che questo può comportare una perdita pari a 2 punti di crescita? Governate dal 2001, da quasi otto anni. Ma vi siete domandati se sarà anche vostra la responsabilità della condizione di questo Paese? Ancora una volta sprecate tutte le occasioni, parlate di sferzata all'economia proponete un decreto che è un guazzabuglio di norme, alcune magari anche utili, ma senza alcuna idea chiara su come, anche attraverso un provvedimento parziale, si possano aggredire le questioni serie di questo Paese. Le misure previste sono poche e scarsamente incisive. Non c'è nulla sulla concorrenza, come ha già detto il collega Agostini e come ha ripetuto il collega Tomaselli. La norma sulla soglia degli appalti sembra essere del tutto discutibile sotto questo profilo, oltre che censurabile per quanto attiene alla trasparenza e alla corruzione. Non c'è niente sul mercato del lavoro e non c'è nulla sulle liberalizzazioni, di cui vi eravate vi eravate fatti paladini; non c'è nulla sul merito e sulla competitività dei talenti. Su questo ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere per la grave situazione del Paese. Come potete pensare che si possa rispondere al tema dei talenti, delle competenze e del merito con questa fantomatica fondazione che avete pensato? Come potete non pensare di avere di fronte migliaia di giovani e di talenti, che emigrano da Sud a Nord, in Europa e se necessario nel mondo, cercando di collocare la loro capacità e la loro competenza in un'attività lavorativa (non certo per scelta)? Questi talenti sono stati formati in Italia; questi talenti sono stati formati grazie a risorse che tutti i cittadini hanno contribuito a mettere in campo, che le famiglie hanno contribuito a mettere in campo, grazie a tanti sacrifici. Questi talenti vanno via dall'Italia; altri si scoraggiano, si arrangiano, si dequalificano, non possono sposarsi, non possono fare figli, non possono progettare il loro futuro. Altro che attenzione alla famiglia e alla natalità! Ma chi l'ha mai visto, da parte di questo Governo, un confronto serio e serrato su questi problemi, la ricerca di soluzioni difficili, ma possibili? A questo provvedimento manca ed è mancata una cosa: la capacità di compiere scelte adeguate e all'altezza dei tempi. È mancato e oggi si esaurisce anche la forza per governare questo Paese. Per tali motivi, anche con questo voto, non avrete la nostra fiducia, sicuri ormai di interpretare un sentimento e un pensiero diffusi in gran parte dell'Italia. Signor Presidente, mi rivolgo al rappresentante del Governo

Pisanu, che sollecita la sua stessa maggioranza e il presidente Bossi a lanciare all'opposizione una sfida per la manovra, per i conti economici e per lo sviluppo del Paese. Il presidente Pisanu dice: lanciamo questa sfida alle opposizioni, vediamo se sono in grado di raccoglierla e vediamo se con loro possiamo assumere le decisioni strategiche del Paese, perché diversamente assumere decisioni in campo economico e finanziario a colpi di maggioranza potrebbe anche insospettire i mercati, facendo apparire il nostro Paese più debole.

quando, nel firmare il provvedimento sulla manovra, ha sostanzialmente detto: auspico che in Parlamento si svolga un confronto realmente aperto, che parta dalla condivisione dell'impegno assunto in sede europea per il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014. Il presidente Napolitano prosegue dicendo di auspicare una seria discussione, libere scelte

alcune misure (come è già stato ricordato dagli interventi che mi hanno preceduto) che sulla carta potevano essere anche molto interessanti, ma che sicuramente, con l'aiuto del dibattito e anche con l'accoglimento di alcune proposte dell'opposizione, che credo non siano sempre da da buttare via, avrebbero potuto essere migliorate. Le faccio due esempi rispetto ad alcuni emendamenti che il Gruppo dell'Italia dei Valori aveva presentato, e che ovviamente

in questo caso con il voto fiducia il lavoro delle opposizioni diventa praticamente inutile; cogliamo tuttavia l'occasione di questi pochi minuti che abbiamo a disposizione prima del voto di fiducia per cercare di far capire agli italiani quali erano le proposte migliorative del testo del decreto sviluppo che come Gruppo dell'Italia dei Valori avevamo presentato. E vengo ai due casi concreti che per brevità tratterò. Mi riferisco in particolare all'articolo 1 del provvedimento in esame, che istituisce in via sperimentale, per il biennio 2011-2012, un credito d'imposta per le imprese che finanzino progetti di ricerca realizzati da università o enti pubblici di ricerca. Credo che puntare sul credito d'imposta per gli investimenti

- riteniamo che, così come è stato scritto il provvedimento, la misura non sembri essere un credito di imposta automatico al 100 per cento. Vi è infatti un sostanziale problema di copertura finanziaria, che sconterà nel tempo l'esigenza di ulteriori verifiche, sino anche a comportare l'eventuale riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. È quindi una copertura assolutamente insufficiente, che rende di fatto questa misura - che, ripeto, sulla carta era interessante - ancora una volta uno *spot* di questo Governo più che una misura di sostanza. Il secondo esempio che desidero portare al Sottosegretario riguarda l'articolo 8, in particolare il comma 5, nella parte in cui modifica la disciplina in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Voglio ricordare che la norma, così come è stata scritta, ha suscitato diversi interrogativi, e non dagli estremisti dell'Italia dei Valori, bensì dalle associazioni rappresentative del mondo industriale, che hanno anche rammostrato la loro difficoltà e le loro critiche rispetto a questo provvedimento. Queste hanno visto nel provvedimento, per come è stato scritto, un'indebita invasione da parte del Ministero dell'economia nelle competenze del Ministero dello sviluppo economico, nonché ancora una volta, com'è abitudine di questo Governo, una sorta di delega in bianco, tesa a stravolgere la missione e le modalità di funzionamento del Fondo. Anche rispetto a questo, il Gruppo dell'Italia dei Valori aveva presentato alcuni emendamenti (ricordiamo che quello dei pagamenti e dei ritardi della pubblica amministrazione è un tema che si trascina da tempo ed è peraltro peraltro di assoluta attualità). Ebbene, avevamo presentato alcuni emendamenti che recavano l'istituzione, in consonanza a quanto previsto nel decreto sviluppo, del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e disposizioni in materia di cessione dei crediti alla Cassa depositi e prestiti; poi, con un altro emendamento, avevamo proposto l'introduzione di una norma, norma, contenuta peraltro nella nostra proposta di contromanovra presentata alla stampa la scorsa settimana, che anche in questo caso recava la cessione automatica alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Provvedimenti quindi che avrebbero potuto incidere positivamente sul decreto sviluppo, ma soprattutto sugli utilizzatori finali di queste norme, che poi sono la nostra linfa vitale: i nostri imprenditori, le piccole e medie imprese, che più di tutte soffrono della crisi economica che sta attraversando il nostro Paese e in particolare, in questo caso, dei ritardi della pubblica amministrazione. Concludo, signor Presidente, signor Sottosegretario, con una sollecitazione, anche se so che rimarrà nell'aria, nell'etere, e non verrà assolutamente accolta: il Governo ripensi seriamente a questa sua modalità di azione. di fiducia su provvedimenti che interessano tutto il Paese, e che quindi dovrebbero essere anche concertati e concordati con le opposizioni, che sicuramente hanno importanti cose da dire, non è un bel messaggio né per il Paese né per l'economia, ma soprattutto ha un solo significato: il Governo Berlusconi si ritrova, ed è in grado di mantenersi in piedi in questa legislatura, *una tantum*, quando vota le fiducie. Dopo di che dimostra - le scorse settimane ne sono state l'esempio eclatante - che quando non c'è il momento della fiducia spesso e volentieri va sotto nei numeri. Quindi, questo significa che c'è una disaffezione da parte dei suoi stessi parlamentari e una poca fiducia nell'azione del Governo. Credo quindi che questo Governo, se vuole dimostrare di avere anche i numeri nelle Aule parlamentari, lo dovrebbe fare tutti i giorni su tutti i voti e non solo su quelli di fiducia.

su un disegno di legge denominato per la promozione dello sviluppo, proprio nell'imminenza della discussione qui al Senato sulla manovra finanziaria necessaria per conseguire l'obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio

signor Sottosegretario, fondato sulla consapevolezza che ovviamente un intervento restrittivo come quello necessario per conseguire al 2014 il pareggio di bilancio strutturale, ha un effetto recessivo sulla economia. Sarebbe meglio dire che avrà un effetto recessivo sull'economia quando, al 2014, la restrizione sul versante della finanza pubblica si determinerà effettivamente, cioè quando, per le decisioni che stiamo per prendere la prossima settimana, dall'economia italiana una quantità variabile tra i 40 ed i 47 miliardi di euro sarà sottratta al fine di conseguire l'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio. Ho detto in altra sede che la consapevolezza del carattere recessivo di una manovra di questo tipo in nessun modo ci deve spingere a considerarla non necessaria: la manovra è necessaria, perché le conseguenze che si determinerebbero sul mercato dei capitali, e quindi sul mercato al quale dobbiamo approvvigionarci per finanziare il nostro debito pubblico, se la manovra non si facesse e se l'obiettivo di medio termine non venisse conseguito determinerebbero sull'economia italiana, sia strettamente dal punto di vista dell'efficienza economica, sia dal punto di vista della giustizia sociale, conseguenze ancor più negative. Ma detto che la manovra è necessaria e consapevoli che ha carattere recessivo,

sul versante della promozione e della crescita che fosse in grado, al 2015 e successivi, di compensare gli effetti recessivi indubitabili che la manovra avrà. Questo è il disegno di politica economica che avrebbe dovuto essere presentato dal Governo e sul quale avremmo dovuto confrontarci. Non è un caso che lo stesso titolo del nostro provvedimento faccia riferimento al semestre europeo: questo decreto sviluppo avrebbe dovuto collocarsi coerentemente nel disegno del nuovo coordinamento della politica economica e fiscale che si sta realizzando dopo la grande recessione in Europa. Europa. Dobbiamo chiederci, responsabilmente, se sia possibile, almeno in linea teorica, individuare interventi di promozione dello sviluppo che nell'orizzonte pluriennale di cui stiamo parlando (2015-2016) abbiano effettivamente la capacità di compensare, sul terreno della maggiore crescita, l'effetto recessivo che certamente la manovra restrittiva di finanza pubblica determinerà.

da adottare immediatamente per la promozione dello sviluppo, per fare in modo di porre in essere subito quelle che, attuate, negli anni che verranno saranno in grado di di determinare quell'effetto di promozione dello sviluppo indispensabile a compensare gli effetti negativi della manovra. È

per non pagare immediatamente il dazio politico ed elettorale che si deve pagare quando si adottano misure restrittive. Questa è una stupidaggine. L'orizzonte pluriennale è indispensabile se si vuole avere lo spazio temporale necessario per adottare misure che, per avere l'effetto economico che ci si aspetta, hanno bisogno di tempo. Certamente conosceremo l'effetto recessivo della manovra di cui stiamo per discutere nel 2014 e negli soltanto nel 2015 e nel 2016 possiamo già stimare che il prodotto interno lordo del Paese, a causa della manovra e

Di cosa avremmo dovuto discutere, quindi, affrontando il decreto sviluppo? Avremmo dovuto discutere di misure che, adottate immediatamente,

come il progresso tecnologico, il livello di formazione del capitale umano, l'efficienza della pubblica amministrazione, del sistema della mobilità, e così via. Se vogliamo che negli anni 2015-2016 - come immagino vogliamo tutti l'effetto recessivo della manovra (che dobbiamo adottare per altre ragioni, altrimenti andiamo a gambe all'aria sul versante della stabilità della finanza pubblica e del sistema Italia nel suo complesso, nel quadro della cosiddetta crisi del debito sovrano dei Paesi europei)

decreto, discutere e approvare misure che agiscano sul versante del miglioramento della produttività totale dei fattori. totale dei fattori dipende da come funziona la macchina pubblica. Il funzionamento tragico del sistema della giustizia civile in Italia deprime gravemente la produttività totale dei fattori.

da Milano a Napoli in otto anni e adesso non riusciamo a completare questa Salerno‑Reggio Calabria, che sembra una maledizione del Paese, la maledizione di Montezuma.

Le misure da adottare su questo versante sono, per esempio, l'apertura della rete del gas. L'Italia va a gas e, quale che fosse la nostra opinione

e potrebbe diventare, attraverso la connessione europea delle reti, l'*hub* europeo del gas. Siamo il Paese in Europa che ha il prezzo del gas più alto, pur essendo collocati geograficamente in modo perfetto per diventare l'*hub* europeo del gas, perché non c'è la separazione proprietaria tra il gestore, un grande campione nazionale, e la rete: l'ENI è, di fatto, proprietario anche della rete, sia pure attraverso la mediazione di SNAM-Rete gas.

Non c'è una grande elaborazione da fare. Certo, c'è da scontrarsi con gli interessi materiali, ben organizzati e molto potenti, soprattutto nel rapporto con la politica, del grande campione nazionale che si chiama ENI; ma, a parte questo, non c'è altra difficoltà. Vogliamo adottare misure che aumentino la produttività totale dei fattori? Questa è forse quella più rilevante, perché ci consentirebbe di pagare di meno il gas; poi, magari, se riuscissimo a fare qualche rigassificatore per approfittare dell'abbassamento del prezzo

Liberazione delle forze più dinamiche del Paese. La produttività totale dei fattori vuol dire questo: liberare le forze più dinamiche del Paese (sia dal lato dei datori di lavoro che dal lato dei lavoratori) dalla persecuzione burocratica cui sono sottoposte, cosicché non riescono a sprigionare la loro potenza produttrice a causa di questa oppressione burocratica (il provvedimento di cui stiamo discutendo avrebbe dovuto essere la sede naturale per fare tale operazione). E ancora, e soprattutto, concorrenza. Ho appena finito di parlare di concorrenza per quanto riguarda le infrastrutture della rete del gas, potremmo parlarne con altrettanta tranquillità a proposito del sistema bancario. Vedo che nella manovra abbiamo messo di nuovo un aumento dell'IRAP, eccetera, e continuiamo a inseguire cose di questo tipo.

sono andati ad esaminare qual è lo *spread* tra gli interessi attivi riconosciuti all'acquirente delle loro obbligazioni da parte delle banche quando fanno un'emissione di titoli verso investitori istituzionali e quando invece fanno emissione di titoli che vengono venduti ai loro clienti. Sapete cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che quando l'emissione ha per riferimento il cliente della banca, in pieno conflitto di interessi, gli interessi attivi riconosciuti sono di un punto percentuale in meno (con il livello dei tassi

La stima è la seguente: a carico di questi risparmiatori abbiamo un aggravio, per mera mancanza di regolazione, di 4 miliardi di euro. I risparmiatori italiani perdono 4 miliardi di euro perché non siamo capaci di fare una regola di una riga che stabilisca che in conflitto di interesse le banche non possono operare, perché non si può essere emettitore di un'obbligazione e venditore di quella stessa obbligazione sul mercato presso il cliente, che si reca allo sportello inerme e che per questa ragione viene espropriato

ed è il punto che riguarda la ricerca, perché il credito d'imposta automatico per la ricerca è una buona scelta, anche se, signor Presidente e signor Sottosegretario (e ne abbiamo discusso in Commissione), l'avete fatto con una tecnica che è è veramente molto grave, in quanto penalizza quelle imprese del quarto capitalismo italiano che sono quelle che ci hanno tenuto in piedi e che vanno sui mercati internazionali, che la ricerca l'hanno fatta anche nel 2008 e nel 2009. Con il meccanismo che vi siete inventati, queste imprese che hanno fatto la ricerca negli anni scorsi, malgrado le difficoltà, verranno penalizzate, perché voi date loro il 90 per cento di credito d'imposta sulla differenza tra quello che faranno in investimenti o ricerca e quello che hanno fatto. Se hanno fatto tanto e continueranno a fare tanto, non prenderanno niente; se invece non hanno fatto niente e adesso faranno qualcosa, prenderanno troppo. È una misura giusta, ma è del tutto squilibrata, e dovreste correggerla. Mi auguro che la correggerete quando ci sarà modo di farlo,

su una questione siamo tutti d'accordo. Le imprese, che hanno il contingentamento del credito, quando vanno in banca non riescono più ad avere i soldi perché le banche non sono in grado, impegnate come sono nella patrimonializzazione, di dare loro i soldi necessari; sono anche taglieggiate dal fatto che lo Stato, le pubbliche amministrazioni le fanno lavorare e poi non le pagano. Il fenomeno dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione è una piaga drammatica nell'attuale sistema economico italiano.

facciamo invece fare a Cassa depositi e prestiti un'operazione attraverso una società veicolo che consenta alle imprese di avere una quota rilevante di quello che debbono avere dallo Stato attraverso questo meccanismo. Ci avete detto di no per l'ennesima volta. Però abbiamo approvato in Commissione un ordine del giorno sul quale, signor Sottosegretario, vi inchioderemo durante la manovra. La La misura che proponiamo noi non è sufficiente, non è corretta, non è tecnicamente ben definita? Trovatene una migliore, ma almeno diamo un segnale a queste imprese, che sono quelle che si sono comportate onestamente. Nel VI secolo avanti Cristo, Solone (l'alleviamento dei pesi) e disse che non può essere ridotto in schiavitù un soggetto che non paga i suoi debiti; deve essere chiamato a rispondere per altri aspetti, ma non può diventare schiavo (ecco perché si chiama *seisachtheia*, l'attività di scuotimento per far cadere giù i debiti). Attraverso quella misura riconobbe libertà

in realtà la base per un'operazione che ha poi portato alla fiorente democrazia ateniese. In Italia, per quello che riguarda le imprese, lo Stato sta dicendo: tu impresa devi lavorare per me, devi essere in grado di stare sul mercato, ma poi io non ti pago e ti condanno a non esistere, a non poter esistere perché non ti pago. È una situazione inaccettabile, di fronte alla quale ci vuole un nuovo Solone, ma dubito che voi possiate esserlo. *(Applausi

Signor Presidente, continuare a parlare della riduzione del numero dei parlamentari e non avviare nemmeno la discussione in Commissione ci umilia e contribuisce a questa decadenza dell'onore della politica e dei parlamentari. In questo senso le sarei molto grato se volesse chiedere al presidente Schifani di sollecitare l'inizio della discussione in Commissione. *(Applausi

come è noto alla Presidenza e all'Assemblea, il 30 giugno è scaduto il decreto di proroga delle missioni militari all'estero. Noi abbiamo pazientato qualche giorno prima di sollevare il problema, anche perché ieri era convocato il Consiglio supremo di difesa, che aveva all'ordine del giorno proprio la razionalizzazione delle nostre missioni militari all'estero. Le agenzie di stampa informano però che in queste ore il Consiglio dei ministri, che era convocato per le ore 9 di questa mattina, non si è ancora riunito perché sarebbe in corso un vertice di maggioranza,

Al di là delle considerazioni di schieramento, è del tutto evidente che i nostri militari, impegnati in missioni ad alto rischio e di grandissima delicatezza politica, si trovano alle spalle un Governo che non è in grado di esprimere un orientamento chiaro su un tema come questo; quindi questo è un aspetto politico di enorme rilevanza. Ma c'è una questione istituzionale: non è immaginabile che si possano tenere i nostri militari all'estero senza un chiaro mandato del Parlamento. Chiedo quindi alla Presidenza di attivarsi perché questo punto sia chiarito in tempi brevi all'Aula e alle forze politiche. *(Applausi

senatore D'Ubaldo.

ci obbliga semplicemente a lasciare una testimonianza attorno ai nodi politici, che rimangono inalterati anche dopo questo dibattito e questo ennesimo provvedimento, il quale dovrebbe ascriversi nella logica dell'avvio e della ripresa dello sviluppo nel nostro Paese. Le condizioni generali sono state oggi politicamente illustrate in un'intervista dal collega Pisanu, il quale invita non solo la maggioranza ma anche l'opposizione a concordare un'operazione di largo respiro per cercare di convergere negli ultimi due anni di legislatura attorno alle scelte strategiche che dovremo pur compiere. Di fronte all'appello del collega Pisanu,

parlamentare e di affrontare il rapporto con l'opposizione, credo che il primo problema sia quello di mettere d'accordo il senatore Grillo con il senatore Pisanu. Nel merito sono state evidenziate tutte le cose possibili ed immaginabili; Commissione abbiamo affrontato il complesso dell'articolato e per ogni punto sono emersi - come sempre avviene attraverso gli emendamenti - gli aspetti critici. A me piace recuperare per *flash* alcune questioni.

che ha centralizzato in capo all'Agenzia delle entrate e quindi ad Equitalia la funzione della riscossione coattiva. Oggi assistiamo ad una tendenziale smobilitazione che metterà in difficoltà per l'ennesima volta e su un altro versante i Comuni italiani. Si tratta di comprendere la strategia, se cioè il Governo ha un'idea generale, oppure

un'azione che non è nell'ordine della trasparenza e della correttezza nei confronti del Parlamento, perché si rappresenta una situazione che non corrisponde alla realtà: in sostanza, si tende ad affermare che una grande ipotesi di lavoro come quella dell'unificazione di due documenti così importanti nella vita del cittadino - progetto su cui si discute da molti anni possa essere risolta attraverso un *maquillage* prodotto con la norma inserita in questo provvedimento. In realtà, ci sono difficoltà che non vengono rappresentate al Parlamento, non vengono discusse in questa sede, non vengono affrontate con serietà, ma che sono presenti e oggettive. Sono due documenti molto diversi: uno è un documento d'identità con la foto della persona, e che serve a circolare, non soltanto in Italia, l'altro è un documento senza la foto, ma con un semplice codice di riferimento. La carta sanitaria viene inviata per posta a tutti i cittadini italiani, mentre la carta d'identità bisogna

Pensare che sia solo un problema tecnico e tecnologico, per cui noi avremmo fatto, con questa norma, un provvedimento che finalmente consenta al Governo Berlusconi di dire al Paese che unifichiamo queste due realtà ben diverse è demagogia

Non è vero che, su un terreno pubblico, non intervenendo una definizione da parte dell'autorità locale si possa fare ciò che immagina il senatore Grillo. Intanto, però, si trasmette questo messaggio. Si riduce la concorrenza,

è evidente che al progetto preliminare accedono solo le grandi aziende. Quindi, si riduce la concorrenza; quindi non stiamo favorendo la competizione per scatenare le energie del Paese, quelle vive, ma stiamo semplicemente compiendo operazioni di natura corporativa. Signor Presidente, concludo il

passaggio dopo passaggio), è solo un messaggio di tipo elettoralistico, ma che non è una risposta di governo a questo Paese. Mi dispiace, e capisco la buona fede e l'intenzione del senatore Pisanu dal punto di vista politico: ma quando mettiamo insieme

a fianco del dibattito esterno e giornalistico, dei *media*, legato alla predisposizione della manovra finanziaria, che è di completa attuazione del Documento di economia e finanza approvato mesi or sono

Documento, che contempla la Decisione di finanza pubblica, la Relazione unificata, il Programma nazionale di riforma ed il Programma di stabilità,

auguro) nel decreto di pubblicazione odierna, che rappresenta il completamento della manovra prevista dal Piano nazionale di riforma e che vedrà impegnato questo ramo

dava un percorso ben preciso e condiviso con l'Unione europea negli indirizzi, nella tempistica e nei contenuti. Sui contenuti possiamo anche

Non viviamo più in un'economia chiusa. Abbiamo un debito pubblico di 1.800 miliardi di euro, il 50 per cento del quale è collocato su investitori internazionali. I tassi dell'economia privata sono strettamente dipendenti dalla credibilità dello Stato. Vorrei ricordare che ieri il rendimento dei nostri titoli di Stato ha superato il 5

quindi uno spostamento di 100 punti base significa 18 miliardi di euro di maggior costo per il bilancio dello Stato. Così vale anche per i tassi interbancari e per il sistema bancario, che ha tenuto durante la crisi. Indipendentemente da ciò che potrebbe essere una aggressione speculativa, dobbiamo tenere i piedi per terra ed essere sempre ancorati alla realtà.

forse peggiori rispetto a quelle economie? Perché ha resistito meglio di altri, pur svantaggiata, alla grande crisi mondiale?

c'era chi voleva che sfondassimo con il debito pubblico. Lo slogan era «aumentiamo il debito pubblico dell'1 come la Spagna di Zapatero». L'esempio della Spagna di Zapatero ce l'abbiamo sott'occhio. Noi non abbiamo fatto come Zapatero; abbiamo sotto controllo i conti, garantiamo il patrimonio degli italiani e abbiamo avuto attenzione per le fasce più deboli. Nel contempo, rispettando i tempi concordati con l'Unione europea, stiamo attuando quanto approvato negli atti di indirizzo

in questo decreto, con particolare attenzione al credito d'imposta per il Mezzogiorno, così come l'intervento sulle opere pubbliche e sul sistema degli appalti, che non è del tutto risolutivo, ma è un modo per eliminare una serie di lacci e lacciuoli che

la semplificazione è un processo che va portato avanti, non è un atto. Non si semplifica con un semplice atto: si semplifica portando avanti una serie di atti che,

si tratta di preoccupazioni di cui la maggioranza si fa carico. Certamente il meccanismo per pagare le imprese che lavorano per la pubblica amministrazione deve essere una delle preoccupazioni del Governo, ma dobbiamo anche fare i conti con quella che è la disponibilità: per pagare è necessario avere i fondi. E la nostra realtà ci porta anche a dover risolvere una serie di altre questioni, quale quella dei Comuni e degli enti locali che possiedono le risorse e che non possono pagare per il Patto di stabilità,

l'Unione europea ci impone. Infatti, su questi vincoli, dai quali non è possibile sforare, si basa il quadro generale. Quindi, il decreto sviluppo è una prima risposta, non è la risposta esaustiva. È cauta, È cauta, forse prudente: può essere forse giudicata troppo prudente, troppo cauta, troppo legata ai conti, ma dà un'immagine del nostro Paese anche di fermezza. E la fermezza sui contenuti

delle Commissioni 5a e 6a riunite senza cedimenti politici di alcun Gruppo di questa maggioranza. Siamo in presenza, quindi, di un provvedimento che ha avuto ampia discussione

i mercati in questi giorni sa che 100 punti di divario nel cosiddetto *spread* fra i rendimenti dei *Bund* tedeschi e dei nostri titoli di Stato ci costano 16 miliardi l'anno» (in realtà un po' di più: 17-18). «E che gli speculatori sono in agguato. Allora sì, che saranno dolori: per noi ma anche per l'euro. Perché l'Italia, con tutto il rispetto, non è la Grecia». Proprio perché siamo maggioranza e sentiamo *in toto* la responsabilità di non manifestare debolezze, che non sarebbero solo nostre, ma del nostro Paese e investirebbero anche l'euro nel contesto internazionale, accogliamo e difendiamo la scelta del Governo di porre la questione di fiducia sul documento in questione. apre una nuova finestra"). Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo. Onorevoli colleghi, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto si svolgeranno in diretta televisiva a partire dalle ore 12. Sospendo pertanto la seduta fino a tale ora.

se ripercorriamo a ritroso le manovre di politica economica di questi tre anni di legislatura, francamente emerge un gigantesco mistero aritmetico. Ricordo, signor Presidente, che abbiamo fatto sei manovre e tre frustate allo sviluppo. Le sei manovre coincidono con le tre manovre triennali più o meno varate tra giugno e luglio, come faremo la prossima settimana, poi ratificate dalla legge di stabilità a dicembre, e su queste si sono sovrapposte altrettante manovre sotto il titolo "decreto milleproroghe": una volta perché si incorporava il gettito dello scudo del rientro dei capitali, un'altra volta per altre motivazioni; ma sostanzialmente si è trattato di sei manovre. Le tre frustate allo sviluppo sono cominciate con la rottamazione dei motorini. Un paio di mesi fa è saltata all'attenzione dell'opinione pubblica l'idea geniale il compito della politica economica è tenere sotto controllo il deficit perché la crescita sarebbe stata garantita dalla modifica dell'articolo 41 della Costituzione. Più recentemente, quattro o cinque giorni fa, stessa musica: compito della politica economica è azzerare il deficit perché la crescita sarà garantita dall'accordo Confindustria-sindacati. Un accordo pregevolissimo e positivo, ma francamente non c'è accordo Confindustria-sindacati che tenga per un Paese che ha il 30 per cento del costo dell'energia elettrica in più, il 15 per cento del costo della logistica in più, e così via. E di chi, se non della politica economica e industriale, è il compito di riforme strutturali e di posizionamento strategico nel settore dell'energia per rendere più competitiva la produzione del nostro Paese?

e qui sta il mistero: avendo già attuato 108 miliardi di interventi, ieri sera all'improvviso, verso le ore 20, appare nel sito del una tabella con i numeri della nuova manovra che dovrebbe arrivare (se non è arrivata stamattina) al Senato, e che discuteremo la prossima settimana, cioè ulteriori 68 miliardi di interventi. ai 51 miliardi di interventi della manovra in quanto tale si sommano all'improvviso 17 miliardi che dovrebbero provenire dalla delega sulla riforma fiscale e del *welfare,* dove in una noticina si dice che o sono maggiori tasse o sono minori spese garantite da una clausola di salvaguardia in automatico. E allora siamo arrivati a 176 miliardi di interventi nell'arco della legislatura. Come mai tutte le manovre effettuate finora determinano oggi un'ulteriore manovra per azzerare il deficit di 68 miliardi? Qui c'è un mistero nel mistero, perché nel recente Documento di economia e finanza era scritto che il deficit nel 2014 sarebbe stato di 46 miliardi: e allora, se c'è da azzerarlo, basterebbe una manovra da 46 miliardi. *(Richiami del Presidente)*. Se invece è di 68, delle due l'una: o il deficit vero non era 46 miliardi, oppure adesso ci proponiamo di avere un avanzo nel 2014 di ben 22 miliardi. Il trucco, signor Presidente (e chiudo sul serio), sta nel fatto che questi tagli sono riferiti ai valori tendenziali degli anni futuri. Nascondono il trucco di mago Merlino: queste manovre per un terzo sono andate a contenere il deficit; per due terzi sono andate a finanziare aumenti di spesa corrente con taglio di investimenti. Allora è evidente che più tasse... La prego di concludere, senatore Baldassarri, perché togliamo spazio alle riprese per gli altri colleghi. che frena la crescita, ricrea deficit e sposta di anno in anno, come una pallina da ping-pong, in avanti il vero risanamento dei conti pubblici. *(Applausi dai

Quando abbiamo letto nel titolo di questo provvedimento le parole «Prime disposizioni urgenti per l'economia» avevamo pensato si trattasse di qualcosa di generale, di strutturale: ma poi, scorgendo via via il testo, ci siamo resi conto che nulla c'era che spostava il carico dei tributi dalle persone e alle cose; nulla c'era che non dico modificasse l'articolo 41 della Costituzione, ma che comunque avesse a che fare con il principio, sempre più invocato e mai praticato, che tutto è possibile, salvo quello che è proibito. Non c'era nulla, perché quelle parole, «Primi», così come tutto il decreto, erano un semplice e demagogico artificio elettorale elettorale nato, consumato e morto al semplice scopo di condizionare e influenzare le ultime elezioni amministrative, successivamente perse rovinosamente da questa maggioranza. Guardate: per quanto ci riguarda, noi non ci sottraiamo alle nostre responsabilità. Se volete, definiamo i saldi che servono al nostro Paese, anche quelli pluriennali, e noi ci impegniamo a rispettarli fino in fondo. Ma in questo decreto non era dei saldi che si parlava, bensì della frustata, della scossa da dare alla nostra economia. Si tratta oggettivamente di un provvedimento modestissimo, fatto da una modestissima maggioranza. Potrebbero essere tanti, gli esempi delle misure sulle quali non siamo d'accordo: sul turismo; sulle sulle poche risorse destinate al credito d'imposta per la ricerca; sulle poche risorse destinate alla detassazione degli investimenti nel Mezzogiorno; sul sistema delle autonomie locali, che stanno esplodendo, e sul il nuovo metodo per la riscossione, non più affidato ad Equitalia, si rischia di creare degli strepitosi buchi di bilancio nei vari municipi della nostra Italia; Grazie ci siamo trovati ad avere a che fare con norme tipo quelle che prevedono l'affidamento senza gara dei contratti di lavoro sotto soglia o l'aumento fino a 1.500.000 euro del limite per gli appalti di lavoro con la procedura ristretta semplificata. esattamente il contrario di quello che, per esempio, sta facendo in questa legislatura Alleanza per l'Italia, presentando norme *ad hoc* che vanno proprio nella direzione di combattere la corruzione che si annida in questo tipo di procedure **(ore 12,08)** (*Segue* BRUNO). Abbiamo presentato altre proposte concrete. Ne cito una su tutte: il taglio dei rimborsi elettorali ai partiti per destinare queste risorse al merito, alla scuola, ai giovani. Ci interessava mettere di fronte, insomma, quel Paese che studia, che si sacrifica e merita, e la cittadella della politica, con la sua possibilità di comprendere una sorta di necessità di partecipare concretamente ai sacrifici generali. Abbiamo presentato norme per provare a semplificare le procedure burocratiche attraverso il sistema dell'autocertificazione alle nostre imprese. Niente da fare: non si riesce a discutere con il Governo e con la maggioranza su come migliorare il modestissimo testo che ci è stato proposto.

necessita e poi, alla prima occasione utile, vi presentate, come al solito, blindati, chiusi, quasi isolati nella vostra maggioranza. Questo provvedimento passerà con il voto di fiducia. Purtroppo per voi, vi allontanerà ancor di più dal Paese reale e farà perdere altro tempo prezioso all'Italia intera. Ed per questo che Alleanza per l'Italia esprime la sua netta contrarietà al provvedimento.

la riflessione già sviluppata sul provvedimento dagli interventi dei colleghi Palmizio, Menardi e Carrara, che ringrazio per il contributo di merito che hanno dato al dibattito, che mi consente di iniziare il mio intervento con una riflessione sull'approccio. Io credo che sia sbagliato, rispetto al provvedimento in esame,

rispetto ad un provvedimento che ha il suo peso, il suo rilievo ed il suo significato, che non può essere banalizzato nella strumentalizzazione del confronto politico. politico. Indubbiamente, infatti, il provvedimento manda dei segnali significativi almeno su tre o quattro questioni. Cito il tema del credito d'imposta per la ricerca scientifica,

e che, come dicevo all'inizio, sia sbagliato l'approccio minimalista da una parte e l'approccio enfatico dall'altra. Noi ci collochiamo, in linea con la riflessione riflessione già sviluppata dai colleghi, in un approccio realista e di consenso critico, citando alcune questioni importanti del provvedimento. A partire dall'articolo 1 e dal credito d'imposta per la ricerca che, a mio avviso, è opportuno mettere in relazione, anche per dare organicità ad alcuni interventi, con l'articolo 9 del provvedimento stesso, cioè con lo strumento del contratto di programma per la ricerca strategica. In questo modo, infatti, ci troviamo di fronte ad un'iniziativa che riguarda il raccordo tra sistema delle imprese, università e centri di eccellenza e tra reti di imprese per la costruzione di contratti di programma capaci di affrontare il tema della ricerca, soprattutto nel Mezzogiorno, come intervento significativo, strutturale e di carattere strategico. Allo stesso modo, riteniamo sia un segnale positivo quello del credito del credito d'imposta per il nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Qui, però, dobbiamo dirci le cose con chiarezza, in relazione sia al credito di imposta per le nuove assunzioni che a quello per gli investimenti nel Mezzogiorno. Signor Presidente, le misure vanno messe in relazione con due questioni. La prima è la copertura di carattere finanziario. Quando la copertura di carattere finanziario riguarda il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo

ma integrativi delle risorse nazionali), da mettere in campo rispetto al riequilibrio territoriale, soprattutto quando tale riequilibrio merita di essere perseguito sul terreno di un deficit che permane e rispetto a spese sia in conto capitale sia in conto corrente squilibrate in maniera

di segnali positivi, ma che vanno concretizzati ulteriormente e che soprattutto nella prossima manovra dovranno trovare elementi di certezza e di concretezza. Non è infatti questo il modo per affrontare e risolvere definitivamente il tema della cosiddetta fiscalità di vantaggio, o fiscalità compensativa, una della leve che il Sud deve recuperare per rendere attrattivi gli investimenti e conseguire la capacità di costruire un modello di sviluppo che vada in direzione della crescita fondamentale non solo del Sud ma dell'intero sistema Paese. Così come sono segnali importanti (e scarsamente attenzionati a mio avviso) quelli relativi

Insomma, c'è un complesso di opere che, se messe insieme a quelle previste dagli articoli 4 e 5 a proposito della riqualificazione delle periferie e degli interventi di semplificazione delle costruzioni, portano a focalizzare l'attenzione su un altro grande tema, tema, quello della cosiddetta leva urbana, che può diventare una leva di crescita e di sviluppo, oltre che di qualità del territorio. Sicché ci sono segnali importanti, positivi, segnali che vanno nella giusta direzione e che debbono trovare ulteriore valorizzazione. A volte, diciamoci la verità, lo stesso centrodestra ha qualche difficoltà a riflettere su quegli aspetti che andrebbero meglio valorizzati anche sul terreno dell'approccio culturale, prima che programmatico, e dell'intervento normativo.

affermato, con grande onestà intellettuale, che oggi il problema fondamentale del Paese e del sistema politico, la domanda cui bisogna rispondere, è come si esce dalla crisi di sistema e si riorganizza la democrazia italiana. Ci troviamo di fronte a una crisi di sistema, e

capacità di dialogo, ma almeno che si recuperi un clima dove innanzitutto possa emergere non solo la responsabilità della maggioranza ma anche dell'opposizione, non fosse altro che per una ragione: sul terreno del grande cambiamento istituzionale e costituzionale l'opposizione ha la responsabilità di avere introdotto una riforma costituzionale il cui impatto non è stato sicuramente utile e funzionale al sistema istituzionale del Paese. Signor Presidente, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, con questa richiesta al Parlamento di un'ennesima fiducia su un provvedimento che pure avevate sbandierato come il vostro cavallo di battaglia per dare una sterzata di sviluppo al nostro Paese, non potete più avere un alibi dietro cui nascondervi: né quello del vostro decisionismo, che non c'è mai stato (nessuno se ne è accorto), un decisionismo che non può attendere le lentezze del Parlamento (dicevate), né quello di un'Europa che chiede scelte e impegni precisi, a cui si deve far fronte con tempi altrettanto certi. certi. Voi sapete benissimo, e lo sa anche l'Europa, che il decreto su cui state chiedendo oggi la fiducia è un provvedimento inutile, confuso, contraddittorio, che non serve alla crescita e non redistribuisce risorse che la prima vera sburocratizzazione di cui avrebbe avuto bisogno il nostro Paese, questa sì a costo zero, è un ritorno alla legalità in tutti i campi. Ora, tutto il Paese ha davanti agli occhi che questo Governo non riesce ad andare avanti se non con la stampella dei colpi di fiducia, che aiutano a tenere incollata una maggioranza che non vuole andare in pensione o, peggio, che sta pensando alla propria pensione. Questo è il triste dato di fatto! Anche se il Governo riesce ancora - e ci auguriamo ancora per poco - a racimolare i numeri alle Camere, non ha più la forza politica di capire e parlare al Paese, di esternare una coesione almeno di facciata, e ha perso ogni residuo di credibilità per poter governare: soprattutto, per governare un Paese come il nostro, che sta vivendo una crisi che mortifica, colpisce e isola i territori e le persone più deboli, il precario che perde il lavoro, le imprese che chiudono, le famiglie che hanno perso la capacità di spesa, di risparmio, di occupazione, il nostro Meridione, che è stanco di aspettare il nuovo annuncio del Piano per il Sud che non verrà mai. Lo dico con tutto il rispetto che bisogna avere nei confronti delle istituzioni: non spetta a noi dire se avete oppure no bisogno di assistenza psichiatrica, come ha suggerito il vostro stesso sottosegretario di Stato alla difesa, l'onorevole Crosetto, perché sappiamo che continuerete sempre a dirci che, in questa crisi internazionale, poteva andare peggio; ma anche al peggio c'è un limite, e voi questo limite lo avete superato, e soprattutto lo avete fatto pesare a tanti italiani. Con le vostre promesse, negli ultimi nove anni del vostro governo, dovevate accrescere per le nostre imprese la produttività e la competitività del sistema Italia: sono entrambe fortemente peggiorate. Dovevate ridurre le disuguaglianze sociali, ma le disuguaglianze sono aumentate. Dovevate riformare una rete di tutela sociale - come aveva detto il ministro Sacconi - che impedisse che la flessibilità del lavoro si trasformasse nell'incertezza del precariato a vita: e questa rete non è stata costruita. Dovevate migliorare i servizi pubblici, statali e locali: ma i servizi sono peggiorati. E non parliamo della riduzione del carico fiscale, riproposta con le varianti una volta al mese da quasi vent'anni: prima, nella sua versione originale, era meno tasse per tutti, poi una riforma fiscale a gettito invariato, oggi una delega a fare la riforma che, quando entrerà in vigore, se entrerà in vigore, troverà le nuove tasse del federalismo fiscale. Dopo gli anni passati a tirare a campare, avete fatto sprofondare il Paese su tre grandi questioni. La prima, economica, perché il vostro non fare a noi italiani costa molto di più del decidere e dell'agire. Nel difficile momento presente, in cui abbiamo davanti a noi la prospettiva di anni di contenimento della spesa e di rigore nelle finanze pubbliche, state facendo perdere al Paese tempo prezioso,

una tassazione delle rendite finanziarie per ridistribuire nuove risorse necessarie a dare respiro alle famiglie e ai soggetti più deboli, un taglio radicale e strutturale dei costi della politica, a patto però che tutto non si riduca al solito *spot* demagogico per prendere in giro l'opinione e la sensibilità dei cittadini.

Da quello che sappiamo dalle anticipazioni sulla nuova manovra finanziaria che ci verrà presentata nei prossimi giorni, riusciamo a capire che l'impostazione di fondo è sempre la stessa, e cioè quella che ha contraddistinto l'azione di questo Governo nei tre anni di legislatura: rimandare gran parte degli interventi necessari al 2013, e scaricare ad altri, sicuramente ad un Governo diverso da questo, ogni genere di responsabilità. È questo il dato di fondo. alla necessità di tagliare - che c'è - un Governo lungimirante individuerebbe le voci improduttive della spesa pubblica, le inefficienze e gli sprechi, che più di altri ci allontanano dall'Europa, e su questo agirebbe con interventi puntuali e mirati. Un Governo debole e diviso, come il vostro, si accontenta invece di andare avanti con blocchi, rinvii e aumenti di tariffe, rimandando gli interventi veri a dopo le elezioni. Per ora agli italiani lasciate i blocchi delle retribuzioni ai lavoratori pubblici, il taglio alle pensioni, i *ticket* sanitari. Veniamo alla seconda grande questione, che è politica: il danno che produce al Paese l'evanescenza di questa maggioranza. Dietro il finto dibattito sulla impostazione della politica economica di Tremonti, dietro le chiacchiere tra i fautori del rigore e quelli della crescita, c'è una resa dei conti tutta interna alla vostra stessa maggioranza. Tutto si svolge solo sul terreno della lotta del potere tra persone e gruppi tra di loro contrapposti. Questa è la verità che dovete dire agli italiani. La P4 di Bisignani è solo un semplice tassello di questo mosaico. Ora per fortuna non è più in grado di fare danni, danni, ma altri centri di interesse, meno chiassosi e forse più potenti, sono, come in altre occasioni, ancora in campo. Lo stesso scontro tra PdL e Lega sui rifiuti a Napoli è un altro epilogo di queste tensioni, ed è grave, è molto grave che non riusciate a capire che questo scontro non danneggia il sindaco De Magistris, ma la dignità di una città e l'intera credibilità di un Paese.

Questo è l'altro grande aspetto che vogliamo porre all'attenzione del nostro Paese. Gli italiani che vi hanno votato hanno accettato di tutto, perché sono un popolo generoso. Gli italiani che vi hanno votato hanno accettato di tutto, perché sono un popolo generoso. Hanno accettato leggi *ad personam*, invettive contro i giudici, le Ruby e le barzellette, ma ora hanno cominciato ad aprire gli occhi e a tirare le somme. Di fronte ad una manovra economica che Tremonti aveva definito etica, ma che chiede nuovi e pesanti sacrifici a pensionati e lavoratori pubblici, nessun Paese civile avrebbe potuto tollerare che il Capo del Governo, pochi giorni prima di una sentenza di risarcimento a discapito della sua azienda, che segue ad una condanna per corruzione di magistrati, provasse a costruirsi una miserevole via di fuga manipolando, all'insaputa dei suoi Ministri, la manovra economica dello Stato con una norma ad uso personale. Un Capo del Governo che non ha pudore di nulla, che non sa neppure far finta di provare cosa siano la disciplina e l'onore che la nostra Costituzione richiede ai propri rappresentanti del popolo, è pericoloso è pericoloso per se stesso e per l'intera Nazione, perché, se prima era mosso solo dai suoi interessi personali, ora è mosso anche dalla consapevolezza che il suo tempo sta per scadere. Noi del Gruppo Italia dei Valori, con la nostra alternativa di governo, accelereremo le lancette di questo orologio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta ci troviamo ad affrontare una discussione artificiale su un provvedimento che avete blindato con l'ennesimo voto di fiducia. Dietro la scusa di velocizzare tempi di approvazione vi è invece la vostra strutturale difficoltà a governare l'Italia. Lo abbiamo già detto tante volte e lo ripetiamo anche oggi: il vostro Governo è paralizzato e questo stato di inerzia rappresenta il male peggiore per l'Italia. testo del provvedimento come una sorta di bandiera per vincere le elezioni amministrative, per vantarvi nelle piazze e nei vostri telegiornali del "governo del fare". Sappiamo tutti come sono andate a finire le elezioni ed il risultato è direttamente proporzionale alla vostra cultura di governo. In un contesto globale in cui si delinea una timida ripresa, l'Italia resta ancora indietro. Il nostro prodotto interno lordo ristagna insieme alla produzione industriale; i consumi delle famiglie restano modesti; la disoccupazione, giovanile e femminile, non smette di gonfiarsi.

La produzione industriale è ferma a meno 0,1 per cento. Ora ci state per sottoporre il nuovo capolavoro, cioè la manovra con annessa la pseudo-riforma fiscale, che ci porterà - dite voi - al pareggio di bilancio. La correzione dei conti pubblici che il Governo si appresta a fare nel corso delle prossime settimane per rispettare gli impegni europei, causerà un'ulteriore depressione del sistema economico, anche a fronte di una ripresa dell'inflazione; in più, scaricate sul futuro il vero peso dell'intervento. In questi anni, signor Presidente, avete promesso tutto a tutti, ma non vi abbiamo mai sentito ammettere una sola delle vostre tante responsabilità. Per voi, infatti, è sempre colpa di qualcun altro: delle opposizioni, della crisi economica, dei mercati, delle agenzie di *rating*. Chissà che prima o poi non sia colpa anche della Spectre! Di sicuro non abbiamo detto noi che le misure contenute nella prossima manovra «andrebbero analizzate da uno psichiatra»: sono parole pronunciate da un vostro autorevolissimo Sottosegretario. Visto che per analizzarle ci sarà tempo in quest'Aula dalle prossime settimane, soffermiamoci sul contenuto del provvedimento in esame che - ribadisco - avete blindato con l'ennesima fiducia perché temete il voto libero del Parlamento e perché non tenete più la vostra maggioranza tanto siete divisi. Forse vale la pena ricordare a chi ci segue in questo momento che a corollario del decreto-legge sullo sviluppo vi è stata la vicenda tragicomica dello spostamento dei Ministeri al Nord. L'un contro l'altro armati, padani contro romani, avete mandato in scena una pantomima senza precedenti che, come sempre, si è rivelata l'ennesima bolla di sapone. Mentre il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 29 per cento, voi vi siete impiccati ad un dibattito surreale, accapigliandovi su una scellerata ipotesi politica che avrebbe fatto - questa sì - lievitare i costi per lo Stato, con buona pace del federalismo. Ora vi presentate con questo provvedimento che appare tanto inadeguato quanto drammaticamente in ritardo con i tempi, perché non aiuta la crescita e non aiuta lo sviluppo del Paese. Questo provvedimento doveva essere la cosiddetta frustata all'economia, ma le uniche cose che avete frustato sono la pazienza e il buonsenso degli italiani, come sulla vicenda delle concessioni balneari; ma quale Governo, se non uno di dilettanti, si sarebbe infilato in un dibattito come questo, senza capo né coda? Avete promesso a migliaia di imprenditori del settore concessioni per altri 90 anni, ben sapendo che l'Unione europea non ve lo avrebbe mai permesso. Avete venduto fumo a migliaia di famiglie che lavorano nel settore, soltanto per racimolare qualche voto in più e avete rimediato una sonora, l'ennesima, figuraccia; e la proroga, come tutti gli altri *spot* governativi, si è sciolta come neve al sole. Grazie a noi avete cambiato timidamente la rotta sul Mezzogiorno: l'unico aspetto positivo presente in questo decreto-legge, che va realmente incontro ai cittadini e agli imprenditori del Sud, lo abbiamo introdotto noi dell'UDC alla Camera con un emendamento per la detassazione degli investimenti per il Sud. Un provvedimento a favore anche di quelle imprese del Nord che vogliono investire e operare al Sud. Sui fondi FAS, invece, che in questi due anni e mezzo avete saccheggiato come Bancomat per la vostra finanza creativa, avete inventato un meccanismo cervellotico e antimeridionale che renderà complicatissimo l'uso delle risorse. Lo stesso avete dovuto fare con Equitalia e con le piccole e medie imprese; la nostra opposizione responsabile ha fatto breccia, perché voi non siete in grado di distinguere tra famiglie e imprese in difficoltà a causa della crisi e gli evasori cronici che si fanno beffe della vostra politica antievasione. A tal punto vi dichiarate contro la patrimoniale, che ne avete introdotta una, perfida e ingiusta, sui piccoli risparmiatori. E avete tentato di farlo anche per i piccoli debitori che, a differenza di quelli del lodo Mondadori, devono pagare subito perché figli di un Dio minore. Per non parlare della scuola, dove avete condannato alla precarietà a vita quasi 20.000 giovani insegnanti che, grazie a questo provvedimento, non avranno la minima possibilità di stabilizzarsi nel mondo del lavoro. Vedete, cari colleghi, con gli *spot* non si governa, ma voi, ormai da quasi tre anni, non fate altro. Ebbene, ci saremmo aspettati la riduzione delle province o la riforma, quella vera, della giustizia, e non il processo lungo, che interessa soltanto qualcuno. Ci saremmo augurati una ventata di liberalizzazioni, tema che avete sbandierato in campagna elettorale e che avete applicato, solo e con tanta tenacia, alla moltiplicazione dei Sottosegretari. In questi anni, spesso in totale solitudine, abbiamo combattuto la logica, pericolosissima, dei tagli lineari. Abbiamo reclamato a gran voce una politica economica più solidale con le famiglie italiane, vero soggetto debole. Siamo stati, purtroppo, sempre inascoltati. Insomma, cari colleghi, signori del Governo, voi date alla crisi economica del Paese è una manovra che si preannuncia come recessiva, perché continua a tagliare, indiscriminatamente, senza incidere sulle sacche, ancora consistenti, dei privilegi; e, contemporaneamente, contrae la spesa destinata agli investimenti e ad incentivare i consumi e la domanda interna. Mentre concepite questa manovra, che scarica sui Governi futuri il costo più importante dei sacrifici da imporre agli italiani, aumentate la pressione fiscale, facendo mettere agli enti locali le mani nelle tasche dei cittadini e disincentivando la propensione al risparmio delle nostre famiglie. l'unica risposta che sapete dare per aiutare la crescita è questo provvedimento che, presuntuosamente, chiamate decreto sviluppo. È un provvedimento piccolo piccolo, che non consentirà di mettere in moto l'economia del nostro Paese, condannato, da anni di politica inutile, alla bassa crescita e all'assenza di competitività. Non è così che si rimette in moto l'economia e voi, pur di galleggiare, logorati dalle vostre divisioni pubbliche e private, continuate a non governare il Paese.

Due Ministri, impegnati personalmente e direttamente sul fronte dei provvedimenti da assumere per rilanciare la nostra economia, i più esposti quindi sulla manovra economica, la pensano tanto diversamente tra di loro che uno, il Ministro dell'economia, dà del cretino all'altro, il Ministro della funzione pubblica; e il terzo Ministro presente, quello del lavoro, dice di non ascoltarlo neanche. Ma in che mani siamo? Dove dobbiamo andare? Dove volete portarci? E ci chiedete pure la fiducia? Ma fateci il piacere! Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, quando, nel dicembre scorso, il Movimento per le Autonomie ritirò la fiducia all'Esecutivo Berlusconi non lo fece per ragioni afferenti a quel periodo particolarmente confuso, in cui il *gossip* prevaleva sulle ragioni della politica, ma lo fece a ragion veduta, sulla base di una valutazione approfondita, a metà legislatura, di quella che era stata la politica economica e la politica sociale del Governo, in modo particolare quella rivolta al Mezzogiorno e quel disimpegno evidente dalle responsabilità che l'Esecutivo aveva fatto di quei territori già al tempo della campagna elettorale. Noi abbiamo allora verificato come in quei due anni e mezzo non vi fosse stata alcuna iniziativa strutturale e d'intervento per le politiche di coesione e vi fosse stato invece l'utilizzo, assolutamente inaccettabile, delle risorse destinate al Mezzogiorno, per garantire i livelli di benessere delle aree più forti del Paese, e vi fosse stata soprattutto una totale insensibilità, un'incapacità di interlocuzione politica con il nostro Movimento rispetto alla proposte che formulavamo, animati dalla speranza che, prima o dopo, anche la goccia d'acqua riesca a perforare la roccia. I nostri temi erano quelli degli investimenti infrastrutturali strategici per garantire uno sviluppo organico del Paese; erano quelli degli incentivi automatici, il credito d'imposta, per arrivare sino alla fiscalità di vantaggio. Era la richiesta di un intervento pubblico in campo di innovazione e ricerca, perché nel Mezzogiorno, senza l'intervento pubblico su questi temi, il *gap* in campo tecnologico e infrastrutturale rimane incolmabile. Invece così non è accaduto, e noi ne abbiamo tratto delle conclusioni. Quando abbiamo avuto tra le mani questo provvedimento, devo dire, signor Presidente, che onestamente ci siamo sentiti sfidati; ci è sembrata un'occasione in cui il Governo andava a vedere le nostre

condizione di aprire una discussione, di essere oggetto di una verifica seria e rigorosa sulla correttezza dei nostri comportamenti politici. Abbiamo poi letto il provvedimento nel dettaglio; le rubriche erano interessanti, il dettaglio ci ha deluso. Il merito delle proposte è insoddisfacente,

credito d'imposta per l'occupazione per un solo anno è insignificante, due anni per i lavori molto svantaggiati: al massimo della capacità può produrre occupazione per 40.000 giovani, quando lo SVIMEZ dice che negli ultimi dieci anni abbiamo perso 360.000 posti di lavoro nel Sud tra giovani e donne. Il credito d'imposta per gli investimenti, insoddisfacente e lacunoso, non garantisce agli imprenditori meridionali una prospettiva di sviluppo stabile e strutturale su cui costruire davvero gli investimenti importanti delle aziende.

l'ha inventata - ancora oggi è inadempiente rispetto ad una serie di adempimenti di cui è responsabile. Quindi, ovviamente, il risultato sostanziale è l'ennesima Abbiamo pensato che potesse essere il caso di un'attività emendativa, che attorno a queste premesse ed intuizioni, a queste novità, potesse svilupparsi un rafforzamento e un irrobustimento della manovra, garantendo risposte concrete. Anche in questo caso, signori del Governo, la nostra iniziativa è stata completamente inascoltata. non un emendamento è stato accolto; al Senato, per le dinamiche parlamentari che vedono oggi posta la questione di fiducia, il dibattito è strozzato, i nostri emendamenti rimangono carta, documenti di un'iniziativa parlamentare senza sostanza, puro divertimento per gli uffici.

Si tratta di alcune intuizioni interessanti, che valgono però come *spot* propagandistici, perché, forse, è prevalsa la preoccupazione di poter dire qualcosa agli elettori e agli imprenditori del Mezzogiorno. Non cambia però la tendenza di questo Governo, le scelte strutturali e la sostanziale prevalenza degli interessi del Nord del Paese: è lì che vengono allocate le risorse. Allora, rispetto a tutto questo, il giudizio rimane negativo. Questo è un Governo lontano dal Sud, se non addirittura ostile. Noi non possiamo votare il provvedimento e non possiamo concedere fiducia a questo Esecutivo. *(LNP)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, l'argomento del giorno è la manovra finanziaria varata in questi giorni dal Governo per annullare il deficit annuo pubblico nel prossimo triennio e quindi finalmente iniziare a ridurre il nostro debito pubblico, purtroppo molto elevato. Sembra quindi passare come in secondo piano il provvedimento odierno dal titolo: «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», ma giustamente definito brevemente decreto sviluppo. Oggi approviamo un provvedimento che concretamente pone mano ad alcuni problemi molto reali reali che toccano i nostri cittadini, le nostre famiglie e le nostre imprese. È su fatti concreti che verremo e che siamo misurati dai nostri cittadini. È questo un provvedimento che aiuta la nostra economia. Il relatore, senatore Mura, ha ben descritto i tanti interventi previsti; vorrei soffermarmi su alcuni anche perché non accettiamo come Lega la campagna di disinformazione fatta dall'opposizione. Parliamo allora di ricerca scientifica e del credito di imposta previsto per finanziamenti ed investimenti, perché siamo per primi assolutamente convinti dell'importanza per uno sviluppo dei Paese delle eccellenze e dell'alta cultura incontro anche ai nostri giovani ricercatori, che possono trovare nel nostro Paese modalità di intervento, di ricerca, di lavoro e di occupazione), oppure la previsione delle zone a burocrazia zero e i distretti turistici, per ora previsti per le zone di mare o costiere ma ritengo debbano essere estesi alle aree montane, specialmente quelli più disagiate disagiate ed emarginate. Questa è un'altra risposta importante alle nostre imprese per poter investire ed essere competitive sui mercati.

e poi gonfiare i costi con varianti e riserve. Noi qui controlliamo che il costo del personale sia giusto; vogliamo opere pubbliche dal costo corretto e nei tempi di realizzazione regolare. Siamo dalla parte delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini con piena trasparenza; altro che le false accuse dell'opposizione di favorire la cricca! é molto brutto questo modo di fare politica con il sospetto e le ambiguità. Non lo accettiamo. Non è nel nostro carattere e non fa parte del nostro comportamento.

La verità è che quelli che dicono che è finito sono coloro che lo vorrebbero affossare. Invece il federalismo è assolutamente attuale, attivo e continua il suo percorso legislativo di completamento. Ci sono poi i tagli alla burocrazia e la semplificazione fiscale. Ci sono insomma fatti concreti che interessano le comunità locali, le persone coinvolte, chi vive e lavora nel nostro Paese. Mi rivolgo quindi ancora una volta, come in altre occasioni, all'opposizione per dire: chiamate poco o inutile tutto questo ? Questo è un momento in cui abbiamo bisogno, come Paese, di compattezza e determinazione nei cambiamenti e nelle riforme necessarie. Noi siamo assolutamente risoluti e decisi. Abbiamo fatto un patto con i cittadini tre anni fa e non verremo meno, non stiamo venendo meno, ai nostri impegni, che abbiamo confermato ed anche rafforzato recentemente a Pontida. Questo provvedimento e la manovra finanziaria che tra breve qui discuteremo sono la prova tangibile di una risposta vera. Sulla manovra, poi, alcuni dicono che spostiamo la correzione finanziaria nel futuro, oltre il 2013 scadenza naturale di questa legislatura), perché non abbiamo il coraggio di farla con questo Governo. Questo è due volte falso. In primo luogo, perché l'abbiamo fatta con responsabilità anche futura, e non solo guardando - magari - a una nostra

strutturalmente e adeguati quando la correzione dei conti pubblici avrà pieno effetto, dando - così - tutte quelle prospettive di crescita di cui il Paese necessita e di cui ha bisogno. Siamo, quindi, pienamente soddisfatti per quanto fatto e ottenuto, nel segno della fiducia che i cittadini elettori ci hanno dato e a cui rispondiamo con concretezza. Questo Paese si cambia lavorando e non facendo continue polemiche. Crediamo che il Paese abbia bisogna di tutto, tranne che di calunnie, polemiche e risse infinite. I recenti scontri in Val di Susa, con le provocazioni e gli attacchi alle forze dell'ordine, sono una brutta pagina che deve essere chiusa e girata in fretta. Va girata lavorando insieme per cambiare il Paese: lo dobbiamo ai nostri precari, ai nostri figli, alle nostre imprese, alle nostre famiglie, ai nostri giovani e ai nostri anziani. Ai nostri giovani - a loro e al loro futuro - deve andare un particolare pensiero. Spesso li vediamo spaesati e persi, come senza possibilità. Dobbiamo capire che serve oggi un nostro sacrificio per un loro mondo migliore. Lo dobbiamo a chi ci ha dato il voto per riformare e cambiare il Paese in meglio. Lavoriamo, quindi, per rendere questo Paese finalmente moderno. Signor Presidente, dichiaro quindi, con convinzione, il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord alla questione fiducia, per i contenuti e per i fatti positivi che il decreto‑legge contiene.

da parte di un Governo ormai ampiamente sfiduciato da tutti gli italiani. Un Governo che cerca di sopravvivere ad ogni costo; un Governo così vicino ai propri interessi quanto lontano da quelli del Paese. Paese. Questo provvedimento, i suoi contenuti e il modo in cui voi avete affrontato la discussione ne sono l'ultima triste conferma. Poteva essere una buona occasione per adottare alcune misure che, anche a costo zero, avrebbero potuto dare un po' di ossigeno ad un'economia in affanno. Bastava solo un accorgimento: quello di far prevalere, per una volta, una volta soltanto, gli interessi generali del Paese su quelli particolari delle caste varie a cui voi siete ormai legati mani e piedi. È per questa ragione che il Gruppo del Partito Democratico (assumendosi la responsabilità che deve avere una grande forza politica, indipendentemente se al governo o all'opposizione, soprattutto in momenti come questi) ha fatto alcune proposte precise, che avrebbero potuto dare sostegno alla crescita del prodotto interno lordo: accogliendo anche una - una sola - delle nostre proposte, si sarebbe registrato certamente un impatto positivo sulla crescita. Del resto, su questo c'è una differenza radicale tra noi e voi: voi ritenete che si possa abbattere il debito con i tagli e senza curarsi della crescita; noi, al contrario, pensiamo che sia impossibile abbattere il debito pubblico senza sostenere lo sviluppo. Con questo spirito abbiamo fatto le nostre proposte, quelle che qui abbiamo illustrato, prima con il nostro relatore di minoranza, il senatore Agostini, e poi con i tanti colleghi che sono intervenuti, e che ringrazio vi abbiamo detto: quei soldi già stanziati per le opere pubbliche, spendiamoli tutti facendo lavorare le tante imprese italiane, con conseguenze positive per l'occupazione, ma questo, non riducendo la trasparenza degli appalti, anzi rendendoli ancora più chiari, perché in questi mesi che le procedure torbide fanno arricchire le cricche e non realizzano le opere pubbliche. La vostra risposta è stata negativa. Votando quel testo, cento degli appalti sarà affidato senza procedura di evidenza pubblica, sarà aggiudicato ai soliti noti e le opere non si realizzeranno. vi abbiamo fatto notare che tante imprese che hanno fatto lavori non hanno ricevuto i pagamenti dalla pubblica amministrazione e questo ritardo sta provocando crisi aziendali, licenziamenti, fallimenti. L'ammontare di questi crediti è stimato attorno ai 40 miliardi di euro. Vi abbiamo detto: utilizziamo la Cassa depositi e prestiti (che ne ha la possibilità) per anticipare almeno una parte di questi pagamenti. Niente. Infine - voglio confessarlo - a una prima lettura ci avevate persino piacevolmente sorpreso su un punto: la reintroduzione di una misura adottata dal Governo Prodi che voi avete cancellato nella finanziaria del 2008. Mi riferisco al credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e innovazione. Tuttavia, non credendo ai nostri occhi, abbiamo riletto con più attenzione il testo: meno male, perché anche in questo caso non vi siete smentiti. Avete rispolverato un titolo di una misura, ma l'avete resa così complicata da renderla inattuabile; inoltre, abbiamo anche scoperto che al fondo è tutta una finta, perché il credito interviene sulla differenza di quanto investito rispetto all'anno precedente: una miseria. Noi avevamo proposto di recuperarla integralmente, l'ennesimo diniego. Insomma, vi siete asserragliati dietro a una serie di ostinati rifiuti, perché la verità è che temete che qualsiasi apertura di una discussione, anche la più innocua, vi esponga a una crisi di Governo. Ormai basta un alito di vento per mettervi in crisi. crisi. Vi chiedo però, signori della maggioranza, fino a quando si può andare avanti in questo modo e a quale prezzo per l'Italia?

Abbiate il coraggio di riconoscere che la crisi finanziaria ed economica mondiale non spiega da sola questi dati; queste sono le cifre del vostro fallimento di questi anni! Così, dietro il titolo roboante di questo provvedimento, state approvando una montagna di chiacchiere, coperta da una propaganda spregiudicata che non incanta più nessuno, anche perché ciascun italiano ormai vive sulla sua pelle le conseguenze della crisi e non si fa più ammaliare da nessuna sirena. In questo provvedimento non c'è una sola misura tra quelle da voi previste che fa crescere il PIL. Doveva essere Doveva essere la scossa all'economia, invece si sta rivelando il penultimo colpo di grazia, perché l'ultimo è rappresentato dalla manovra che avete appena approvato nel Consiglio dei ministri: una manovra di cui siamo venuti a conoscenza a piccole dosi, come si fa con quei prodotti particolarmente velenosi, con norme annunciate e ritirate nel modo più confuso, con continui distinguo nella maggioranza (ho visto che poche ore fa il ministro Tremonti ha dedicato un pensiero particolarmente gentile al ministro Brunetta) e con quelle anonime manine che appaiono e scompaiono per lanciare i sassi, come è accaduto con il famoso codicillo "ad aziendam". Ci avete fatto assistere per l'ennesima volta a quel consueto modo di fare del nostro Presidente del Consiglio, di chi tira il sasso e nasconde la mano. Un modo di fare che ha raggiunto un tale ritmo in questi tre anni che neanche si può più parlare di sassi, perché quella che abbiamo di fronte ormai è una frana, la fragorosa frana di una politica, di una maggioranza e di un Governo. proprio quando ci sarebbe tanto bisogno di un Governo che sappia impiegare al meglio le risorse di cui è ricca l'Italia, per creare beni pubblici, capitale umano e sociale, un Governo che sappia rompere quel groviglio di compromessi che garantiscono rendite, corporazioni, lavoro nero, esclusione sociale, soprattutto delle nostre donne e dei nostri giovani: di quelle ragazze e di quei ragazzi sui cui progetti di vita ormai pesa come un macigno lo spettro violento e terribile della precarietà. Ecco, proprio in questo momento invece dobbiamo prendere atto della più amara delle realtà: noi siamo un Paese senza una guida, senza una rotta. Un Paese dunque che sta rischiando grosso, e ne abbiamo avuta la conferma nella dura vicenda dei rifiuti di Napoli, quei rifiuti scomparsi per il tempo necessario a celebrare le doti taumaturgiche del Presidente del Consiglio. Come per il terremoto in Abruzzo, quello dei rifiuti doveva essere il trofeo da esibire: è stata la *summa* dei vostri inganni. Sono riapparsi, ancora più di prima, e sotto lo sguardo cinico, egoista e distaccato di una classe dirigente che sta offuscando anche uno dei valori fondamentali che è sempre stato un valore di riferimento nei momenti più difficili degli italiani, quello della solidarietà. Voglio concludere, signor Presidente: il ministro Tremonti ha definito questo decreto «una legge che si legge»: ecco, proprio perché si legge, caro Ministro, questa è una legge che non regge, come non può più reggere questa situazione. Il nostro voto contrario al provvedimento e a questo Governo è da interpretare come l'atto di una forza politica, la nostra, che sente tutto il tutto il peso della responsabilità di chi dovrà restituire un futuro a questo Paese: quel futuro che voi gli state rubando. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, avevamo promesso che avremmo dato un segnale al Paese e oggi iniziamo a mantenere la promessa. Fin qui abbiamo assicurato la stabilità nonostante la più grave crisi economico-finanziaria dal 1929; abbiamo garantito la coesione sociale e la tenuta dei conti del Paese; abbiamo fatto sì che l'Italia, di fronte allo spettro del fallimento di Stati sovrani, si trovasse dalla parte di chi era in grado di aiutare e non fra coloro che avevano bisogno di aiuto. Oggi ci accingiamo ad approvare un provvedimento che fin dal suo nome, decreto sviluppo, segna una ripartenza ed un rilancio. Un rilancio non effimero, perché poggia sulla stabilità e non si nutre di quella spesa in deficit che scaricherebbe il nostro presente sul futuro dei nostri figli. Un rilancio non episodico, non contingente, poiché è solo il primo passo di un percorso che da qui al 2014 porterà l'Italia a pareggiare il proprio bilancio così come non questa maggioranza, ma il Paese intero si è impegnato a fare con l'Europa. Presidente, sarò ingenuo, ma mi ero illuso che al dunque l'opposizione avrebbe messo da parte la propaganda e la strumentalità per scrivere insieme una pagina per il Paese, approvando misure che non si possono non condividere perché agevolano l'impresa, incentivano l'occupazione dei più deboli e lo sviluppo delle aree sottoutilizzate, valorizzano le nostre specificità e puntano a ridurre la distanza fra Nord e Sud; perché allentano le maglie soffocanti di una burocrazia divenuta nei decenni ipertrofica, mettono fine a vessazioni inique, smentiscono la falsa e fuorviante equazione secondo la quale, a procedure più snelle ed efficienti, dovrebbe corrispondere una minore trasparenza. Questo provvedimento dimostra che è vero l'esatto contrario. È tutto ciò che serve? Certamente no, ma è tanto di ciò che in questo frangente storico ci è consentito di fare, anche con un pizzico di fantasia alla quale la limitatezza delle risorse disponibili impone di far ricorso. Eppure, colleghi della sinistra, voi vi opponete oggi a questo provvedimento per lo sviluppo. Lo fate un po' per strumentalità politica e un po' nascondendovi dietro quella singolare professione professione chiamata "benaltrismo" di cui fra le vostre file vi sono alcuni professori emeriti, per la quale di fronte a qualsiasi proposta, invece di valutarla nel merito, si dice che "ben altro" servirebbe al Paese. *(Applausi se è sul metro del "ben altro" che dobbiamo misurare le nostre risposte di Governo, cominciamo col dire che ben altri sono i sacrifici che Paesi civilissimi dell'Occidente hanno imposto ai propri cittadini per far fronte alla crisi. Ben altri sono stati i tagli alla spesa e le strette sui servizi. Ben altre sono state le ricadute in termini di disoccupazione e impoverimento in certi Paesi socialisti dai quali l'opposizione di casa nostra ci ha a lungo invitato a prendere esempio: valga su tutti la Spagna di Zapatero mentre in Italia il Governo e la maggioranza hanno destinato decine di miliardi di euro agli ammortizzatori sociali. Smentitelo, se ne avete la possibilità. Signor Presidente, molti non se ne sono accorti, probabilmente neanche in quest'Aula, ma nel pieno della crisi l'Italia è scesa dal podio nero dei maggiori debiti pubblici del mondo: se prima eravamo al terzo posto, ora la Germania ci ha superato, perché la sua situazione pregressa le ha dato la possibilità di reagire alla crisi aumentando la spesa pubblica. Noi questa opzione non l'abbiamo avuta, nemmeno come possibilità, a causa della zavorra di debito pubblico che grava sulle nostre spalle. Se l'avessimo praticata, per il nostro Paese sarebbe stata la catastrofe. Nel cortile di casa nostra l'opposizione ha preferito non considerare tutto ciò per crogiolarsi sulla scia di recenti e singolari sortite di qualche agenzia di *rating* sulle cui tempistiche e modalità la CONSOB fa bene a chiedere chiarimenti. E allora c'è da chiedersi, e senza retorica: perché la nostra opposizione sembra gioire ogni volta che un'agenzia di *rating* solleva un dubbio per l'Italia e tace quando la stessa agenzia, come è evidenzia rischi per la Spagna, per il Portogallo, per la stessa Francia, mettendoli a confronto con il differente percorso del nostro Paese? Non c'è in questo atteggiamento una sindrome antinazionale *(Applausi dal Gruppo nel modo in cui vengono alimentate campagne denigratorie sui giornali stranieri, manovre di Palazzo e aggressioni mediatico-giudiziarie? In piena coerenza con questo atteggiamento, colleghi della sinistra, oggi dite ancora una volta no, e, quando vi si è chiesto di suggerire qualche alternativa, avete saputo proporre soltanto nuove spese senza copertura. Dovrete spiegarlo agli italiani perché dite no al credito d'imposta per le imprese che finanziano la ricerca, che investono nelle aree sottoutilizzate e che nelle Regioni del Sud assumono lavoratori svantaggiati. Perché dite no a misure che autorizzano l'emissione di titoli di risparmio per l'economia meridionale fiscalmente agevolati

Dovrete spiegare perché dite no a un provvedimento che mette un freno a misure di riscossione coattiva eccessivamente rigide, che rende meno farraginose le detrazioni fiscali e le procedure contabili, che incentiva la riqualificazione urbanistica ed edilizia garantendo al tempo stesso maggiore trasparenza, che interviene sulla pianta organica di settori strategici, che incrementa la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che rende più attrattivi gli investimenti nel nostro Paese, che valorizza le specificità italiane nel settore turistico, portuale ed agricolo. L'unica cosa su cui oggi non dovrete dare spiegazioni, colleghi dell'opposizione, è il vostro voto contrario a misure che rendono più semplice far nascere un'impresa: in questi giorni, infatti, avete dimostrato che voi le imprese preferite farle morire. Per noi, signor Presidente, colleghi senatori, la difesa dell'impresa ha un valore sociale primario perché significa difesa dei lavoratori, delle loro famiglie, dell'avvenire dei loro figli. E lo consideriamo un principio assoluto, indipendentemente da questioni di metodo, di grammatica istituzionale e di galateo; soprattutto, senatore Latorre, è per noi un principio che vale se l'impresa fa riferimento a un nostro amico politico ma vale a maggior ragione se l'impresa è di un nostro avversario. Per questo, signor Presidente, nelle prossime ore insieme al presidente Gasparri e a tutto il Gruppo del PdL presenteremo un disegno di legge che riproponga in termini strutturali e ben articolati quella norma su cui tanto si è polemizzato e che, proprio per via di queste polemiche, è stata eliminata dalla manovra Tremonti appena licenziata dal Governo. Ne parleremo a tempo debito. Crediamo però che tutto questo abbia molto a che fare con l'economia e abbia molto a che fare con lo sviluppo. A proposito dello sviluppo, Presidente, l'Aula si accinge a licenziare un provvedimento importante, che tocca snodi nevralgici dello Stato sociale e del sistema produttivo del Paese. Non siamo così presuntuosi da ritenere che da oggi le difficoltà siano superate. Crediamo però che sia un buon inizio, e che per inseguire il «ben altro» impossibile l'opposizione abbia perso un'occasione per contribuire al rilancio possibile. Noi questa occasione non la vogliamo perdere, ed è per questo che annuncio il voto favorevole del Popolo della Libertà.

Passiamo al voto sull'articolo unico del disegno di legge n. 2791, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.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 ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Hanno chiesto di votare per primi pochissimi

Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Maritati, Mascitelli,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

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: